L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

a conclusione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, colleghi il disegno di legge n. 591, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 10 marzo scorso, il cosiddetto decreto Cutro, muove dai tragici accadimenti del 26 febbraio scorso. La maggioranza di Governo e il Governo hanno impiegato cinquanta giorni per scrivere norme senza adeguati chiarimenti, che non ci sono arrivati nemmeno nelle lunghe giornate trascorse in Commissione, che, proprio alla luce di quei fatti,

rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, per l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Che i flussi migratori verso l'Italia, così come verso tanti altri Paesi d'Europa - e non solo - non siano un'emergenza, ma un fenomeno strutturale, pare evidente alla grande maggioranza di analisti e studiosi e agli esponenti istituzionali. Ne cito uno: il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Zuppi, ha detto che emergenza è un fenomeno molto maggiore di questo. Ancora gravi sono i rilievi che muoviamo alle modifiche che il testo apporta in materia di protezione speciale, che afferiscono al diritto di asilo, e di divieti di espulsione e respingimento, per la complessità degli istituti coinvolti, di cui non si è tenuto conto. Giova qui richiamare l'articolo 10 della Costituzione italiana, secondo cui lo straniero privato delle libertà nel suo Paese «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica». Rileviamo inoltre, davvero con estrema preoccupazione, che, a differenza di quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'interno e da molti altri esponenti della maggioranza e del Governo, il provvedimento in esame non contiene alcuna misura volta a scongiurare il rischio che si ripetano tragedie analoghe a quella di Cutro. È davvero ridicolo, anzi grottesco, associare il provvedimento ai fatti di Cutro. L'articolo 1, che riguarda la programmazione dei flussi legali, prevede che siano assegnate quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovano campagne mediatiche sui rischi dei viaggi in mare. Onorevoli colleghi, è davvero un'assurdità grottesca, più che ridicola, perché non tiene conto della tragica realtà dei fatti e degli eventi internazionali.

Voglio citare il Sud Sudan, che in queste ore ci fa immaginare come dev'essere la qualità della vita di quelle persone, ma anche la Siria, l'Afghanistan e purtroppo tanti altri Paesi. Ebbene, noi immaginiamo che lì vengano fatte campagne mediatiche, per spiegare alle persone che non devono partire? Voglio poi citare l'articolo 2, che dovrebbe recare misure di semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di lavoro, che assegna a categorie di professionisti, togliendola all'Ispettorato nazionale del lavoro, la responsabilità di procedere a tutte le verifiche, come l'asseverazione delle condizioni. Questo avviene in assenza di parametri precisi a cui attenersi, come se esistessero persone di serie A,

Ancora di più ci preoccupa l'articolo 7, che sopprime il divieto di respingimento e di espulsione di una persona, qualora esistano fondati motivi per ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti

del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Quali sono le ragioni di merito, di necessità e di urgenza, secondo l'articolo 77 della Costituzione, per abrogare questa forma di protezione speciale? Davvero non è comprensibile. Il diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E voglio sottolineare che, a differenza di quanto è stato sostenuto proprio in questi giorni dal Governo e dalla stessa Presidente del Consiglio, non è vero che una larga parte dei Paesi dell'Unione europea non preveda e non abbia in vigore norme del tutto simili alla protezione speciale che l'Italia ha Questa possibilità è del resto prevista dalla cosiddetta direttiva rimpatri del 2008, dal Codice frontiere Schengen, dal Regolamento di Dublino e dal codice dei Infine, suscita davvero una grande preoccupazione l'articolo 10, laddove prevede la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri questa sia effettuata fino al 31 dicembre 2025 in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sono

Si tratta di norme che voi calate dall'alto sulla testa dei sindaci e dei presidenti delle Regioni e non soltanto di quelli delle Regioni del centrosinistra. Ascoltate anche i vostri presidenti di Regione, perché saranno loro a essere chiamati a gestire quotidianamente la presenza dei migranti e il loro rapporto con i cittadini. In realtà, non averli ascoltati e rifiutarsi di ascoltarli e di coinvolgerli come bisognava fare dà un'idea davvero molto preoccupante di come voi immaginate la democrazia. Questo intero provvedimento, a ben vedere, è semplicemente ispirato da una logica punitiva nei confronti dei migranti, poco lungimirante e per niente risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, che potrebbe essere solo con una riforma profonda della normativa sugli ingressi, con un sistema di accoglienza solido e con un supporto all'integrazione sociale, alla creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante, perché noi vogliamo che per ogni migrante ci sia una cornice di diritti, ma anche di doveri. Voi rifiutate di fare ciò che serve a questo Paese e lo fate solo per ragioni di consenso, contro i principi di umanità e di saggezza a cui invece dev'essere improntata una riforma

riteniamo questo decreto profondamente incostituzionale. Quello che esamineremo è un decreto - com'è stato adesso ricordato - che nasce all'indomani della strage di Cutro e che però, contrariamente alla dichiarazione di intenti e addirittura contrariamente al nome che un po' indebitamente porta, non contiene a nostro avviso alcuna norma volta ad incidere concretamente per evitare le stragi in mare, nemmeno per limitare le partenze. Viceversa, è un decreto che tradisce una logica totalmente punitiva - con l'intento di colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese - che peraltro mette anche le 10.000 persone che oggi usufruiscono della protezione speciale e già vivono nel nostro Paese in una condizione di grande difficoltà e che certamente rischia di spingerle all'irregolarità. È inoltre un decreto che ha l'obiettivo di smantellare il sistema di secondo livello di accoglienza e integrazione in favore delle misure di prima accoglienza. Questo però non è casuale: evidentemente, avviene perché le misure della cosiddetta prima accoglienza sono meno costose e provvisorie. Soprattutto, sono misure che non prevedono nessun elemento di inclusione dei migranti nel nostro sistema sociale: è come se si volesse dire, in maniera chiara e definitiva, che il migrante viene trattato come un problema e non come una risorsa. Ciò è evidentemente conseguenza di un ragionamento che viene fatto da molto tempo a questa parte, secondo il quale

Riteniamo che il decreto-legge sia incostituzionale perché adottato in violazione dei principi stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Si tratta peraltro di un decreto-legge con più contenuti distinti, il cui testo non è omogeneo; inoltre, sono del tutto carenti i presupposti

si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali e con i principi internazionali in materia di asilo. noi riteniamo in contrasto con la Costituzione e i principi internazionali in materia di diritti fondamentali l'articolo 7, che sostanzialmente sta abrogando la protezione internazionale per motivi familiari, l'articolo 8, che prevede pene spropositate ed equipara condotte molto diverse, in questo caso mettendo clamorosamente in discussione un principio cardine

e anche illustrando i tanti emendamenti che abbiamo presentato e che abbiamo cercato di presentare in Commissione, dopo aver atteso per giorni che la maggioranza risolvesse le divisioni e le contraddizioni che aveva al proprio interno, dal nostro punto di vista l'articolo 7 è la disposizione più critica di tutto il provvedimento: viene abrogato il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale. Non starò a discutere di tutte le questioni più tecniche di modifica della disciplina della protezione speciale, cioè l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1 (poi lascerò agli atti una un testo

si può rilevare in qualunque manuale di diritto pubblico. Per l'appunto, quell'articolo 10, che garantisce il diritto di asilo per lo straniero, viene invece messo radicalmente in discussione nel momento in cui si va a colpire un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario, che è esattamente quello che si sta facendo in questo momento, peraltro - lo devo dire, ma anche questo lo ripeterò

a un dato secondo il quale il nostro Paese sarebbe l'unico in Europa ad avere nell'ordinamento nazionale, oltre alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria (quindi all'asilo),

che accompagnano gli strumenti di protezione internazionale anche con uno strumento di protezione speciale. Sono molti, per l'appunto, i Paesi dell'Unione in cui sono in vigore norme assimilabili a quella che avevamo noi. Peraltro, questa possibilità è prevista espressamente dalla direttiva rimpatri, ma anche dal codice frontiere Schengen e dallo stesso regolamento di Dublino, che pure noi abbiamo mille volte criticato, ma che questa disposizione contiene.

Le disposizioni abrogate dall'articolo 7, invece, rispondevano esattamente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare ed è assolutamente evidente - a me pare che un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di uno straniero tale da costringerlo a rompere il sistema di relazioni sociali e familiari creati all'interno dello Stato ospitante costituisca un'interferenza molto seria nella sua vita privata e familiare.

la clandestinità e anche i migranti che oggi vivono in Italia regolarmente saranno messi in una condizione molto più difficile. Devo dire anche che contestiamo con grande forza

incriminatrici generiche e non tassative e pene non proporzionali alla gravità del fatto. Potrei andare avanti a lungo, perché sono tante le ragioni d'incostituzionalità, anche quelle contenute quelle contenute all'interno dell'articolo 9, laddove si prevede l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni in caso di provvedimenti concernenti il soggiorno: altra cosa incredibile, perché sostanzialmente si nega

per i rimpatri, ci sono evidentemente una serie di anomalie e di elementi molto discutibili, anche perché le locuzioni che vengono utilizzate - a questo è stato fatto riferimento anche nell'intervento precedente della senatrice Zampa - sono talmente vaghe e generiche

lo considero un decreto-legge profondamente anticostituzionale e soprattutto un provvedimento profondamente propagandistico, che non risolverà nemmeno una delle questioni politiche delle quali stiamo discutendo, ma anzi aggraverà profondamente la situazione del Paese.

come voi sapete il Gruppo di Azione-Italia Viva è piuttosto restio a intervenire sulle questioni pregiudiziali d'incostituzionalità. Noi riteniamo che la questione pregiudiziale vada posta con molta parsimonia e oculatezza, solo nei casi in cui sia manifestamente fondato il dubbio d'incostituzionalità di una norma. Ci darete atto in quest'Aula di non aver utilizzato il tema della pregiudiziale per motivi ostruzionistici, anzi; la nostra preoccupazione è che, a furia di gridare sempre «al lupo al lupo» sull'incostituzionalità di una norma, poi possa succedere che non ci accorgiamo con la dovuta attenzione quando una legge è realmente fuori dalla cornice di legalità costituzionale. Oggi, però, sentiamo il dovere d'intervenire sul punto della costituzionalità. In questo mio intervento mi limiterò ai profili più strettamente giuridici, mentre in discussione generale entrerò più nel merito della questione dal punto di vista politico. Faccio una doverosa premessa: questa norma, il disegno di legge n. 591, di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, per me non si chiama e non si chiamerà

per rispetto di quelle persone che hanno trovato la morte al largo di Steccato di Cutro e per le 390 vittime che sono state ritrovate morte nel Mediterraneo nei primi tre mesi di questo 2023. Non chiamatelo decreto-legge Non chiamatelo nemmeno decreto immigrazione, perché le norme, peraltro in parte condivisibili e di buonsenso sulla programmazione triennale dei flussi, sulle semplificazioni e sull'accelerazione delle procedure, sono solo la prima parte di un *corpus* normativo che stiamo analizzando oggi. Come si chiama allora questo decreto-legge che oggi ci troviamo a convertire? Per me si chiama decreto-legge sicurezza-*ter*. Perché? Anzi tutto, perché risponde a una logica securitaria, non di governo dei flussi migratori, ed è il terzo provvedimento che si affianca al n. 113 del 2018, anche noto come decreto-legge sicurezza - che rappresentava la politica migratoria dell'allora ministro dell'interno Salvini - e al decreto sicurezza-*bis*, il n. 53 del 2019, che si occupava invece del fronte esterno.

due rilievi: ma come? Avevate promesso agli italiani che con voi al Governo la pacchia per i migranti sarebbe finita e non siete riusciti nemmeno a fermare una - e dico una sola - delle imbarcazioni dai porti di partenza?

Dov'è l'invasione dei tartari alle nostre porte? Evitiamo di raccontare balle agli italiani. Nel 2022 sono giunte in Italia attraverso il Mar Mediterraneo 105.000 persone; nel primo trimestre del 2023 sono già arrivate 20.000 persone, con un aumento del 320 per cento. Come dimostrano i numeri, la vostra presenza al Governo non è affatto un deterrente per l'arrivo dei migranti in Italia tant'è vero che il Ministro dell'interno, riprendendo le parole del presidente della CEI, ha detto che non esiste in Italia alcun allarme; esiste uno stato d'emergenza tecnicamente inteso. Sono parole del Ministro dell'interno, quindi smettiamola di usare termini impropri: non esiste alcun allarme invasione migranti; non esiste alcuna emergenza migratoria. L'unica vera drammatica emergenza del nostro Paese si chiama demografia, si chiama denatalità e a questa rischia di aggiungersene un'altra grave, che si chiama ignoranza, quando un Ministro della Repubblica, parlando d'immigrazione, evoca persino la sostituzione etnica. Non credo che queste espressioni vengano utilizzate per motivi razziali, né per motivi suprematisti. Credo invece che lo si faccia per ignoranza, nel senso di ignorare non quello che dicono i senatori in Aula, ma quello che dice il DEF. *(Applausi)*. Tale documento afferma che per andare avanti in alcuni settori dell'economia italiana ci vogliono flussi migratori. Eccola, l'ignoranza. però non ci arrendiamo all'ignoranza, alla propaganda vuota dei porti chiusi e a quella - mi dispiace dirlo anche agli amici dell'opposizione - di un'altrettanto vuota retorica dell'accoglienza, per cui diciamo "venite, c'è posto per tutti, tanto poi vi facciamo passare dall'Italia e il problema lo scarichiamo agli altri Paesi europei". No, la retorica dei porti aperti e dei porti chiusi è il vero motivo per cui da decenni non governiamo i flussi migratori, ma usiamo la questione migratoria per mero consenso politico. Torniamo alla legge in esame. Non esistono i presupposti di necessità e urgenza di questa decretazione semplicemente perché non c'è alcun allarme di invasione dello straniero. È illegittima la decretazione d'urgenza che introduce fattispecie incriminatrici e tecnicamente inopportuna altresì l'idea di procedere con emendamenti e subemendamenti, anche di rilievo penale, per modificare una norma che è già entrata in vigore al tempo dell'emanazione del decreto. Fin qui il metodo, ma andiamo al merito. Sono almeno tre i profili di forte dubbio di legittimità costituzionale. Mi soffermo sul primo: la soppressione della protezione speciale. Facciamo un passo indietro. La protezione dello straniero in Italia si fondava prima del 2018 su tre pilastri: lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Nel 2018 il Governo Conte I emanava il decreto sicurezza, su impulso dell'allora ministro Salvini, per eliminare la protezione umanitaria. Raccogliendo le formulazioni della Presidenza della Repubblica sulla base della giurisprudenza costituzionale e in conformità al diritto dell'Unione europea e agli obblighi internazionali, il ministro dell'interno Lamorgese, nell'allora Governo Conte II, emanava il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, configurando una forma di protezione speciale che di fatto ripristinava l'istituto della protezione umanitaria nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute. Che cosa vuole fare il Governo oggi? Vuole abolire la protezione speciale. Perché lo vuole fare? Le considerazioni politiche sono due. La prima: è un *unicum* in Europa. La seconda: è attrattiva dell'immigrazione illegale clandestina. Andiamo a vederle. È un *unicum*? No, come ha già rilevato il mio collega De Cristofaro. Tale misura esiste nella maggior parte dei Paesi europei, solo che non si chiama protezione speciale, ma protezione per motivi umanitari. è attrattiva dell'immigrazione illegale? Andiamo a vedere i numeri. Secondo le stime approssimative, in Italia ci sono circa un milione di migranti irregolari o clandestini. Sapete quanti sono coloro che hanno beneficiato della protezione speciale? Quanti sono? Un milione? 100.000? Quanti sono? Sono 10.865 casi. Allora, colleghi senatori, non siamo davanti a un *unicum* italiano, né davanti a un fattore attrattivo dell'immigrazione. Il problema semmai è un altro.

invece di migliorare il sistema dell'accoglienza, nel senso che vi dirò dopo, nel secondo intervento, avete scelto la scorciatoia di tagliare la protezione speciale, in spregio alle norme costituzionali, all'articolo 10,

fermatevi, voi che potete, davanti al rischio d'infrangere la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale. Ragionate sul fatto che i flussi migratori non si fermano davanti alla deterrenza della norma, perché non c'è paura di una legge che possa mai essere superiore alla paura di morire.

cancella la parte del testo unico sull'immigrazione che disciplina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Sappiamo bene, invece, che l'articolo 10 della Costituzione, al terzo comma, garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo recependo il diritto europeo in materia di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario integrato dal sistema d'asilo. Contrariamente a quanto dice il Governo e in particolare la presidente Meloni, la protezione speciale trova fondamento anche nell'ordinamento europeo, specialmente nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riguarda esattamente il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare. Sulla base di queste norme, la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento dello straniero dal territorio degli Stati parte della Convenzione. I permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti anche dalla direttiva europea n. 115 del 2008, si legge: «In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare Corte di cassazione, a partire dalla sentenza n. 4455 del 2018, nel fare riferimento alla vita privata e familiare, ha riconosciuto la rilevanza dell'integrazione sociale per quanto concerne l'accertamento di condizioni di vulnerabilità che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria. Sembra quindi che nella visione del Governo la declinazione dell'articolo 8 della CEDU non possa essere riconosciuta nell'ambito della protezione speciale nazionale, stante l'abrogazione che viene fatta dell'esplicito richiamo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Così non è e neppure può essere perché il complesso normativo sull'immigrazione è quello che ho appena detto. In definitiva, il testo previsto dall'articolo 7 del decreto quindi non solo si pone in contrasto con i nostri principi costituzionali cui all'articolo 10 della Costituzione, ma pone l'Italia inadempiente nei confronti non solo della giurisprudenza interna, ma anche di quella della Corte Europea dei diritti umani, ora ad alcune considerazioni di tipo politico. Le disposizioni del provvedimento sono di mero stampo propagandistico: non solo violano il diritto nazionale ed europeo, come ho appena dimostrato, ma nemmeno perseguono lo scopo dichiarato, che sarebbe quello di ridurre gli sbarchi. La protezione speciale non ha nulla a che vedere con gli sbarchi e con il loro numero e la maggioranza, inclusa la presidente Meloni, lo sa benissimo. Partiamo dai numeri, che sono stati da poco ricordati. Nel 2022 sono stati rilasciati 10.865 permessi di protezione speciale: il 36 per cento è stato concesso a cittadini albanesi; il 24 per cento a cittadini peruviani; a seguire, a persone provenienti dal Mali. Come vedete, i due Stati maggioritari non hanno nulla a che vedere con gli sbarchi: le persone non arrivano via mare. Ricordo - e lo sottolineo - che l'intera America Latina è stata esclusa dal decreto flussi, che giustamente non chiamiamo decreto Cutro. queste persone non hanno nulla a che vedere con gli arrivi dal mare: sono persone già integrate in Italia e che spesso lavorano nel settore dei servizi alla persona, sostanzialmente come badanti. coloro che, per capirci, accudiscono i nostri anziani, di cui pure vi riempite la bocca. Voi li gettate nell'irregolarità, fate perdere loro il lavoro e ai nostri anziani la persona di fiducia. si farà, quindi? Si pagheranno in nero o si manderanno via? Questa è la scelta di fronte a cui si troveranno i datori di lavoro di queste persone che voi additate come illegali, mentre siete voi a renderli tali con questo provvedimento. Ancora una volta, state perseguendo misure vuote, buone per nascondere la vostra totale incapacità di agire sotto una cortina fumogena di propaganda. Raccontate all'opinione pubblica che la protezione speciale non esiste in Europa e che porta i migranti a scegliere l'Italia perché qui da noi c'è, quando quando invece sono ben diciotto i Paesi dell'Unione europea in cui è prevista una protezione simile alla nostra, e in molti di tali Paesi coloro che godono di questo tipo di protezione sono assai di più di coloro a cui è riconosciuta qui in Italia. evidente che negare ad alcune persone il diritto a vedersi riconosciuto il rispetto della vita privata e familiare, dell'effettivo inserimento sociale in Italia e dei legami culturali, sociali e affettivi significa

In una parola, si chiama disumanizzazione *(Applausi)*, che è la precondizione necessaria alla discriminazione e al fomentare l'odio. Come si spiegano altrimenti le ripugnanti parole del vostro ministro Lollobrigida, che parla di sostituzione etnica, con un linguaggio che va al di là di ogni misura tollerabile? E non è ignoranza, lo ribadisco: ormai lo schema è chiaro e noi del MoVimento 5 Stelle non ci cadiamo. Tutti i giornali oggi parlano del disappunto della *Premier*, perché la sua classe dirigente, con queste continue uscite, irricevibili in un consesso civile, disfa di notte la credibilità la credibilità che ella cerca di tessere di giorno. Balle, sono balle. La *premier* Giorgia Meloni è nata e cresciuta in quello stesso brodo di coltura in cui sono nati e cresciuti tutti i Lollobrigida del partito di maggioranza. Loro dicono semplicemente ciò che lei non può più dire. Vergogna. Per raccattare qualche voto in più non vale la pena alimentare odio e frizioni sociali, calpestare il diritto nazionale e internazionale, isolare il nostro Paese a livello europeo e gettare nell'illegalità - quindi nel mercato nero, se va bene, o nelle maglie della criminalità organizzata, quando va male - decine di migliaia di persone,

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è già stato detto che l'esame di questo provvedimento dovrebbe interrompersi. Abbiamo presentato a tale scopo la questione pregiudiziale e riteniamo che esso sia completamente sbagliato, per tutta una serie di ragioni che cercherò di illustrare. Siamo molto dispiaciuti di dover affrontare nuovamente l'argomento del governo dei flussi migratori un grande fenomeno strutturale del nostro tempo - a partire da un provvedimento che non si pone affatto lo scopo di migliorare il governo dei flussi migratori, ma soltanto di trovare la maniera per strumentalizzarli politicamente nel modo nel modo che, ad avviso della maggioranza, è più efficace per la sua convenienza immediata. *(Applausi)*. Questo è avvenuto con il decreto-legge che sostanzialmente aveva la finalità di complicare la vita alle organizzazioni non governative che salvano le vite in mare; questo avviene con il decreto-legge improvvidamente ribattezzato "Cutro". "Cutro". Dico improvvidamente perché a Cutro è avvenuta una grande tragedia umanitaria e invece le tracce di umanità nelle disposizioni di questo provvedimento sono difficilmente ravvisabili. È un provvedimento che si presenta doppiamente prigioniero. In primo luogo, prigioniero di un dissidio nella maggioranza: infatti, una parte della maggioranza ha bisogno di sventolare un vessillo e di dire che con questo provvedimento si torna al passato glorioso dei decreti Salvini; e un'altra parte della maggioranza, invece, che esprime la Presidenza del Consiglio, spesso ha avuto una propaganda consonante con quella dei decreti Salvini. In virtù delle responsabilità che copre attualmente, però, sa che insistere su quel percorso porterebbe al nostro Paese più danni che vantaggi, ma da questa prigionia non riesce a emanciparsi. La confusione di questi giorni è il frutto di questo contrasto insanabile di punti di vista e di interessi. Poi, tutta la maggioranza in generale è prigioniera - e questa è la seconda prigionia

che avevate fatto dall'opposizione è concretamente attuabile e realizzabile, vi scontrate con questo dato di fatto e non sapete come cavarvi d'impaccio. Da qui i pasticci, gli errori e le scelte molto gravi sul piano dei valori. Questo provvedimento è un fallimento. È un fallimento sul piano del merito, è un fallimento sul piano del metodo, è un fallimento sul piano dei valori. Lo è sul piano del merito per quattro ragioni, che cito rapidamente. La prima è l'idea che si debba colpire il sistema dell'accoglienza diffusa: è una sciocchezza, questa. Il sistema dell'accoglienza diffusa va rafforzato, non colpito. Il secondo errore è quello di decidere di credere alla fola, alla falsità che l'esistenza della protezione speciale, così come esiste nel nostro Paese dal 2020, sia un fattore che alimenta le partenze verso il nostro Paese e attrae flussi migratori. Questo è falso. Dovreste smettere di dirlo e dovreste anche smettere di crederlo: per il vostro bene, per il nostro bene e per il bene del Paese. Ciò vi porta a creare infatti una situazione nella quale

l'evidente contrasto con le norme del diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la nostra Costituzione. Questo lo sapete, perché l'ossessione del ritorno ai decreti Salvini è l'ossessione del ritorno a provvedimenti che hanno subito la sorte che conosciamo. Tali provvedimenti sono stati demoliti e derisi da giuristi italiani ed esteri, sono stati oggetto di obiezioni formali del Capo dello Stato in sede di promulgazione infine, in punti non secondari, sono stati rasi al suolo da pronunciamenti della Corte costituzionale. Sapete quindi che un giorno questo provvedimento arriverà di fronte alla suprema Corte di legittimità costituzionale le parti evidentemente in contrasto con il diritto europeo, con le convenzioni internazionali e con la Costituzione non sopravvivranno. A voi però non interessa che sopravvivano, perché a quel punto avranno già raggiunto già raggiunto il loro scopo: aver creato la percezione che, finalmente, c'è chi esibisce i muscoli, fa la faccia feroce e sa essere molto duro contro deboli e disperati che non possono difendersi. Non è un gran lavoro dovreste provarne un po' di vergogna. *(Applausi)*. Sul piano del metodo, quello che avete fatto non va bene, perché, per portare avanti questa campagna propagandistica, avete deciso di chiudervi al confronto con i Gruppi di minoranza in Parlamento. Non abbiamo avuto modo di veder approvato nessun nostro emendamento, nemmeno emendamenti che erano palesemente ragionevoli e approvabili, non animati da alcun intento ostruzionistico. Vi siete chiusi al confronto con l'associazionismo più impegnato nell'integrazione e nel soccorso a queste persone disperate, associazionismo che ieri ha protestato in piazza della Madonna di Loreto e davanti ai palazzi del Senato, in maniera molto ferma. Avete deciso di essere sordi a tutte queste obiezioni, a tutte queste rimostranze e a tutte queste proteste; soprattutto, avete deciso di celebrare una rottura con il sistema delle Regioni e degli enti locali, senza il quale nessuna integrazione seria è possibile nel nostro Paese. però - e vado a concludere - tutto quello che sto dicendo non vi tange, perché non avete l'obiettivo di fare un'integrazione seria. Credo che debba essere detto in maniera molto chiara che l'obiettivo che state perseguendo è quello di portare avanti quella che potremmo chiamare una nuova politica della tensione: alzare la tensione su un problema per racimolare qualche consenso, disinteressandosi del fatto che, invece di risolvere i problemi, se ne creano di nuovi. Qui veniamo al fallimento sul piano dei valori. Insomma, con le scelte che avete compiuto abbiamo un dibattito pubblico su questo argomento che è meno civile e meno umano, che è stato immiserito da queste forzature e che è diventato più meschino e più gretto. A tal proposito - e finisco davvero - vorrei dire qualche parola in merito a ciò che è avvenuto ieri. Io ieri mi sono vergognato come cittadino di questo Paese, mi sono profondamente vergognato di fronte alle dichiarazioni del ministro Lollobrigida. E vorrei che - come me - pronunciasse parole di vergogna la diretta superiore del ministro Lollobrigida, cioè la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che da queste dichiarazioni non trarrà alcun beneficio. Perché mi sono vergognato? Mi sono vergognato per il contenuto delle dichiarazioni: la teoria della sostituzione etnica è una teoria di chiarissimo conio e stampo razzista, antisemita, cospirazionista e suprematista *(Applausi)* e non dovrebbe avere nessun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico italiano nel 2023.

è stata fatta da un Ministro della Repubblica italiana nel giorno stesso in cui il Capo dello Stato ha pronunciato parole indimenticabili ad Auschwitz *(Applausi)*, dove il razzismo e l'antisemitismo hanno prodotto i guasti più grossi. Il nostro Paese da questi fatti esce screditato, si isola, è meno credibile nel portare avanti azioni per stringere alleanze a livello internazionale, che sono l'unico strumento con il quale possiamo pensare di fare un salto di qualità nel governo dei flussi migratori possiamo pensare - altro che alla sostituzione etnica! - alle cose che sono scritte nel DEF firmato dal ministro Giorgetti, che ci parla della necessità, per soddisfare le esigenze delle imprese e delle famiglie italiane, di fare una buona integrazione di centinaia di migliaia di lavoratori nei prossimi decenni. E allora avremmo bisogno di canali legali per l'inserimento il più possibile calibrato sulle esigenze delle famiglie e delle imprese. Di questo dovremmo discutere; dovremmo interrompere la politica della tensione e avviare una buona politica dell'integrazione. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto ringrazio il mio Capogruppo e gli altri Capigruppo di maggioranza, che mi hanno delegato a fare questo intervento in merito alle due questioni pregiudiziali sulle quali l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi. Tali questioni pregiudiziali sono una plastica rappresentazione dell'atteggiamento che, come abbiamo visto, in questi giorni è stato tenuto dalle opposizioni, soprattutto da alcune di esse, in Commissione affari costituzionali,

in uno in modo assai scarno e con poche righe, in un altro in modo più argomentato, vengono poste questioni squisitamente di merito, relative semmai al dibattito che ci sarà.

Come dicevo, però, ciò è del tutto coerente con l'atteggiamento e la linea che abbiamo visto in questi giorni, nei quali, in Commissione affari costituzionali, le opposizioni - in particolar modo il Partito Democratico, la sinistra - hanno ritenuto di esercitare un vero e proprio ostruzionismo, che in questa prima fase di legislatura, in Senato, non si era visto a questo livello sicuramente di uno strumento legittimo della dinamica parlamentare e democratica, ma dobbiamo evidenziare che in questo caso viene utilizzato da partiti che hanno tutti governato e quindi contribuito a determinare la situazione esistente,

anche al fine di evitare tragedie come quella di Cutro e le molte altre che l'hanno preceduta: pensiamo a quella del 2015, al largo del Canale di Sicilia, e a tante alte. La contabilità, forse anche prudenziale, ci parla infatti di oltre 26.000 morti nel Mediterraneo: è una contabilità di guerra. pensiamo che non vi sia nessuna contraddizione tra questi due elementi cardine del decreto-legge, perché non contrastare l'immigrazione irregolare significa delegare agli scafisti e ai loro criminali mandanti la gestione dei flussi migratori. A questo proposito, è emblematico anche quanto emerso ieri su alcuni *media*, in relazione a un video girato da presunti scafisti, che, con lo sprezzo di chi lucra sulla vita dei migranti, spacciavano la traversata quasi per un viaggio comodo e tranquillo. Questo ci dice quanto la volontà di spezzare il filo del traffico di esseri umani sia la strada giusta. Questo è l'impegno che dobbiamo alle vittime di Cutro e di altre tragedie simili. In questo modo le possiamo onorare, non certo con le ignobili manifestazioni con i *peluche* contro il Governo, che corrispondono solo a una categoria: quella dello sciacallaggio politico. contrasto all'immigrazione illegale, dicevamo, serve anche per organizzare meglio quella legale, perché è vero che abbiamo bisogno anche di lavoratori stranieri, ma, come accade in tutta Europa e in tutti i Paesi industrializzati del mondo, dobbiamo poter individuare i settori e le specializzazioni necessarie, nell'agricoltura, nell'industria, nel turismo e in tutte le categorie e i settori che hanno queste necessità. Ecco perché vogliamo che sia chiaro agli italiani che, in un momento storico in cui la crisi in Tunisia, un Paese che aveva una linea di fermezza e di collaborazione rispetto ai traffici d'immigrazione illegale, che oggi vive una fase d'instabilità, si aggiunge al fronte libico già aperto per quanto riguarda gli ingressi illegali dalla fascia subsahariana, la sinistra, anche con queste questioni pregiudiziali, si oppone, come non aveva mai fatto in sei mesi, a un decreto-legge che vuole introdurre un nuovo reato per colpire duramente i responsabili della perdita di vite umane. Caro senatore Parrini - mi rivolgo al Presidente, ma rispondendo a quanto ho sentito lei si vergogna delle dichiarazioni di un Ministro che stava semplicemente dicendo che ben vengano i flussi migratori regolati e la buona immigrazione, ma che si vuole anche promuovere l'occupazione femminile che è a livelli bassissimi

decreto, che voi non volete neanche si ponga in discussione,

per i Paesi che fanno campagne per disincentivare le partenze? Volete cioè che non vengano disincentivate le partenze dei barconi sui quali le persone perdono la vita? Forse pensate che non siano sufficienti, ma perché non volete queste campagne? Anche su questo ci dovete rispondere.

che, specialmente in seguito al decreto dell'ex ministro Lamorgese, ne hanno fatto una sorta di *escamotage* per una sanatoria permanente. Dobbiamo ricordare che la protezione speciale riguarda principalmente i cittadini che vengono da Paesi definiti sicuri e non

divieto di espulsione da utilizzare solo in casi delimitati e inoppugnabili, ad esempio a fronte del rischio d'induzione al matrimonio forzato e negli altri casi previsti dalla norma. si tratta solo di cavilli che hanno alimentato false speranze nei migranti, hanno paralizzato gli uffici dello Stato e hanno determinato degrado e insicurezza nelle nostre città. A questo proposito, ho letto che alcuni sindaci del PD si sono svegliati e hanno paventato il rischio tendopoli. Noi vorremmo far loro sommessamente notare - io vengo da una lunga esperienza di amministratore a Roma e posso parlare per la mia città tendopoli e bivacchi li abbiamo spesso e continuativamente visti. Basta farsi una passeggiata al Tiburtino, alla stazione Termini, al rione Esquilino, a piazza Vittorio, così come in tante piazze d'Italia nelle quali abbiamo la plastica rappresentazione del modello che voi volete difendere. Ci accusate quindi di legare sempre il tema della sicurezza all'immigrazione e ci dite anche che abbiamo una fissazione securitaria, quasi evocando una maggioranza che vuole imporre uno Stato di polizia, ma noi vi ricordiamo che se c'è quest'associazione è proprio perché un modello fallimentare ha portato le persone, oggi, ad avere paura a tornare a casa la sera. E ciò accade perché qualcuno, quando ha governato, ha detto che bisognava aprire indiscriminatamente le porte a tutti e ora anche dall'opposizione vorrebbe imporci questo modello. *(Applausi)*. Ora però ci siamo noi

gestita tenendo conto delle proprie necessità, e a un forte contrasto all'immigrazione illegale, anche a tutela di coloro i quali mettono a repentaglio la propria vita affidandosi a mercanti di uomini ai quali noi non daremo mai tregua.

recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

non ha potuto concludere le votazioni riguardanti tutti gli emendamenti e i subemendamenti che erano stati presentati. Nonostante abbiamo lavorato a lungo

intorno a questo provvedimento si è costruita una narrazione che talvolta poco ha a che fare con quanto esso prevede realmente. Questo decreto-legge - lo ricordava prima il collega de Priamo e sono contento di intervenire dopo di lui, proprio per dare un *continuum* a quanto stiamo raccontando stabilisce numeri certi per i comparti di cui abbiamo necessità per i flussi migratori. Estende inoltre la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a tre anni invece che a due, com'era precedentemente, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. Pone poi attenzione - di questo si è parlato poco

i vostri giudizi su tutto ciò che concerne questo aspetto e soprattutto su chi, come queste persone, molte volte ha la responsabilità delle tante morti che abbiamo subito nel Mediterraneo? C'è l'articolo che sopprime l'intimazione a lasciare il territorio entro giorni: anche di questo abbiamo parlato poco, perché questa è una misura che ci chiede l'Unione europea. Parliamo dell'Unione europea solo quando fa comodo a qualcuno? Quando invece l'Unione europea ci dice cose sulle quali poi il Governo interviene, anche per dare maggiore sicurezza e certezza a queste misure, facciamo finta di niente. C'è conseguentemente la misura che prevede il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri. C'è poi la madre di tutte le battaglie, quella di cui si è parlato costantemente, come se fosse il tema di quello che dovrà avvenire in futuro, cioè il tema della protezione speciale. Voglio ribadire ancora una volta quello che già è stato detto da molti: ovviamente non stiamo togliendo obblighi europei e internazionali - ci mancherebbe - che prevedono già tante forme di protezione, tutte quelle che garantiscono a una persona che è davvero a rischio di vita e di discriminazione di non dover essere rimpatriata. C'è poi la protezione speciale, sulla quale pure talvolta abbiamo sentito delle inesattezze, delle inesattezze, perché è un caso *unicum* in Europa per quello che riguarda il nostro Paese e perché siamo stati gli unici ad attivarla. Ci sono solo altri quattro Paesi in Europa che hanno attivato un processo particolare, tra cui la Spagna, che però ha un elenco specifico di fattispecie su cui questa protezione può essere attivata, tra l'altro dall'azione di un magistrato, che deve prevedere che si entri all'interno di tale fattispecie; c'è poi la Germania,

mentre le domande di asilo e delle altre protezioni sono cresciute solo del 76 per cento. Vi rendete conto di quale differenza stiamo ponendo in essere? Voglio dirlo con una certa chiarezza i numeri anche qui parlano chiaro: sapete qual è la nazionalità che è stata maggiormente premiata da questa protezione? La comunità albanese, per il 36 colleghi che sono in quest'Aula ieri hanno partecipato alla riunione congiunta delle due Commissioni delle politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, dov'è venuta a trovarci la Presidente della Commissione integrazione europea del Parlamento albanese. Cari colleghi, vi sembra un Paese da cui bisogna scappare? Vi sembra un Paese - per quello che ci è stato raccontato - in cui c'è questa grandissima necessità di protezione? Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di una misura che evidentemente allarga i confini di un'immigrazione che, di fatto, è molto lontana da quello di cui si parla. L'Italia allora, in realtà, con questo decreto-legge ha compiuto il primo passo di una strategia più complessiva sul tema dell'immigrazione, perché questo è un altro fatto che va sottolineato con chiarezza. Abbiamo posto questo tema nei confronti dell'Unione europea, e lo sapete perché lo abbiamo detto, lo abbiamo ascoltato anche dal nostro Presidente del Consiglio: per la prima volta l'Unione europea ha posto il tema dell'immigrazione come uno degli obiettivi da poter raggiungere nei prossimi anni. Ne stiamo parlando proprio per capire come un fenomeno

per dare un destino diverso ai Paesi dell'Africa e quindi anche per risolvere il problema dell'immigrazione. Concludo, Presidente, dicendo che non ci arrenderemo all'idea che uomini, donne e bambini possano rischiare la vita in viaggi della speranza per poi essere abbandonati nelle nostre città senza integrazione e senza aiuto, pensando che tutto questo si chiami solidarietà. Non ci arrenderemo all'idea che si possa abbandonare l'Africa e si possa e si debba per forza vivere lontano da quel Continente, come dicevano due persone di spiccato profilo, una

Su questo lavoriamo, proprio perché sappiamo che il vero conflitto è tra chi pensa che ci sia una visione di fluidità che non prevede confini, appartenenze e tradizioni. Noi siamo per l'identità della persona, di genere. Ci piacciono le identità locali e nazionali; capiamo e vogliamo riscoprire il senso di comunità proprie radici e non ci arrenderemo a non raccontare la bellezza e la forza di queste idee.

questa è la vicenda politica, il succo politico della questione. Volete mettere una bandierina, che non riuscirà a fermare i flussi migratori perché, come dicevo prima, non sono né la deterrenza né la paura della legge a poter fermare la paura di morire. Nel primo intervento ho detto che l'abolizione della protezione speciale non è altro che un modo in cui di fatto si vuole ritornare con le lancette al 2018, quando si era abolita la protezione umanitaria. Ho detto che non va bene il sistema dei porti chiusi, semplicemente perché anche voi avete dimostrato, con la vostra presenza e con l'aumento del 320 per cento, che i porti non saranno mai chiusi, e non va bene il principio dei porti aperti, soprattutto quando diciamo: passate e il problema e il problema se lo gestiranno gli altri Paesi europei. Il nostro dovere è dire piuttosto come si governano i flussi migratori. Si governano su tre pilastri: lavoro, sistema di accoglienza e cooperazione internazionale. Per quanto concerne il lavoro, qual è l'errore che state facendo? Aumentare la programmazione da due a tre anni? Certo che va bene, ma, signori, avete mai conosciuto qualcuno che assume una persona al buio? Assumereste mai una persona al buio? Potete pretendere o chiedere che i nostri imprenditori assumano persone che non hanno mai visto? *(Applausi)*. Lo volete capire che un sistema d'inserimento lavorativo si fa con la formazione mirata, non sulla base di numeri? Stiamo parlando di persone, non di pacchi. Smettete di avere un approccio logistico, quando si parla di persone. il sistema di accoglienza ci sono tre passaggi di questa catena: gli *hotspot*, che dovrebbero funzionare da sistemi d'identificazione; i CAS, che dovrebbero funzionare da sistemi di centro di accoglienza straordinaria; il SAI, che dovrebbe essere il fulcro di questo sistema di accoglienza e integrazione. La nostra logica è che l'attenzione dovrebbe essere concentrata tutta sul SAI, che ricade sui Comuni. *(Applausi)*. Invece voi che cosa volete fare? Volete ritornare indietro nella catena, pensando che la parolina magica degli *hotspot* sia il fulcro dal quale gestire il tema dell'accoglienza. Signori, il rischio è che voi trasformiate un centro d'identificazione in un luogo di detenzione informale *(Applausi)*, privando le persone dei diritti e delle libertà fondamentali. È questo l'errore concettuale. Bisogna potenziare il sistema di accoglienza e integrazione e lavorare verso la formazione e l'inserimento lavorativo e invece voi volete tornare indietro, perché perché questo sistema produrrà immigrazione irregolare. Ritorno al punto: creare un problema per avere consenso dal problema creato e non risolverlo, ma sfruttarlo come un'opportunità di crescita ed integrazione per tutti. Altro elemento: la cooperazione internazionale. Se noi fermiamo, tutti quanti, le rotatorie della propaganda cominciamo insieme a pensare che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nel contesto europeo, difenderemo i confini nazionali come europei attraverso una riforma seria del Regolamento di Dublino sulla base del principio di leale cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri. Non potete dire che se ne deve occupare l'Europa, ma poi non le date la competenza affinché se ne possa occupare; sono questi il fraintendimento e l'ipocrisia che ci sono dietro questa situazione. Dobbiamo difendere i confini nazionali perché europei, attribuendo le competenze all'Europa perché li possa esercitare propriamente. È lì che si esercita la sovranità nazionale, non declamandola. Altro elemento: la cooperazione internazionale. Non basta evocare il piano Mattei (poi un giorno ci spiegherete - oltre al nome evocativo del piano, che tutti noi non possiamo che approvare - cosa c'è al suo interno). La cooperazione internazionale si fa cercando di capire un elemento fondamentale: non ci può essere protagonismo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale, se il Mediterraneo, anziché essere un cimitero delle speranze di intere popolazioni, non ridiventa, nella cultura e nella civiltà europea, un luogo di scambio, di crescita, di opportunità di sviluppo e di coesione. Ricordatevi sempre - e con questo concludo - che la mitologia greca, che evidentemente dovrebbe insegnarci qualcosa, raffigurava l'Europa come una donna che attraversava il mare, dal Sud al Nord, per fuggire da una violenza. Questa è l'idea di Europa che noi dovremmo propugnare: una forza gentile che attraversa il mare, dal Sud al Nord, al Nord, per portare pace nel mondo, in Europa e nei nostri Continenti.

Paradossalmente, l'essersi avvicinati al luogo della tragedia ha reso ancor più evidente la distanza tra quel Consiglio dei ministri e quello che succedeva intorno. un decreto-legge che non dà risposte a quella tragedia, né esprime alcuna capacità di governo di un fenomeno strutturale. È un decreto irresponsabile, disumano e, per certi versi, grottesco, come diceva stamattina la senatrice Zampa. Creerà più irregolari, più lavoro nero e nessuna inclusione. Il provvedimento è nato male, appunto, ma l'*iter* è proseguito ancora peggio,

della maggioranza, della vostra maggioranza, di votare in Commissione gli emendamenti del Governo: un fallimento. Eppure, di fronte all'INPS, che ricorda che i migranti salvano le nostre pensioni, di fronte agli schemi del vostro DEF, che dimostrano che i migranti salvano la nostra economia, e di fronte ai dati reali, che prendono il sopravvento sull'ideologia, il nervosismo mette all'opera il solito dispositivo, la logica mai inclusiva, che contrappone i diritti di alcuni a quelli di altri e usa i diritti di una parte contro quelli degli altri. Sfugge l'idea che l'inclusione sia produttrice di benessere per tutti. Adesso il mantra è "prima le donne": non ci provate! *(Applausi)*. Non provate a usarci contro i migranti. Non provate a buttare la palla dell'occupazione femminile per non affrontare questo nodo. Pensate piuttosto a come non far fallire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché lì come Paese ci eravamo dati un obiettivo sull'occupazione femminile, ma ci avete perfino chiesto di stralciare da un ordine del giorno le linee guida sulla clausola del 30 per cento dell'occupazione femminile. Non usate le donne come un esercito di riserva contro quella che voi vedete come un'invasione.

modo in cui il Paese guarda al futuro, al benessere delle donne, al *welfare* e alle politiche per la famiglia, perché poi - ed è questo il punto - al di là dei benefici per il PIL e al di là dei numeri squadernati nei documenti economici, c'è qualcosa che viene prima. Stiamo parlando di persone che fuggono per migliorare la propria vita. Lo voglio dire sommessamente, anzi, neanche tanto: l'umanità è una, nessuno sostituisce qualcun altro. È una vergogna quello che abbiamo sentito ieri dal ministro Lollobrigida *(Applausi)* e aspettiamo le scuse della presidente Meloni. Ci siamo vergognati: sono complotti usati dalla peggiore destra nel mondo quelli che pensano alla sostituzione etnica. In ogni caso, tutte le motivazioni di questo decreto si basano su cose non vere: emergenza, invasione, gli unici ad avere la protezione speciale. La storia e la realtà ci dimostrano che i flussi migratori non sono arrestabili e che non cessano le ragioni umane, politiche ed economiche che spingono le persone a rischiare la vita per lasciare i propri Paesi. L'Europa e l'Italia hanno il dovere di adottare una legislazione utile, come ha ricordato in Polonia il presidente Mattarella. Fermatevi,

una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale, con grande senso di responsabilità. Quello che chiediamo all'Europa - perché è giusto chiederle di cambiare - dobbiamo chiederlo a livello nazionale. Servono progetti per la formazione e l'inserimento lavorativo:

Abbiamo di fronte persone. Il problema è creato dall'incapacità di programmazione e di governo di questo fenomeno strutturale. [**Presidenza ma poi il vostro ministro Piantedosi ci ha spiegato, di fronte ai rilievi della CEI, che questa emergenza è uno strumento tecnico per adottare provvedimenti veloci ed efficaci. Quindi «non esiste un allarme, ma esiste uno stato di emergenza tecnicamente inteso»: così ha detto il Ministro. C'è pertanto un uso strumentale dei poteri di emergenza e, per ciò stesso, illegittimo. Il sottosegretario Molteni ancora ieri in Commissione ha voluto sottolineare che non si deroga sui diritti, ma sulle procedure. Eppure la chiusura totale verso i nostri emendamenti, verso quelli che mettevano in prima linea una maggiore garanzia sui diritti, non solo ci fa permanere il dubbio, ma ci dà conferma. Insisto: fermatevi; fermiamoci e facciamo un piano nazionale. Se anche il Ministro riconosce che non c'è emergenza, ascoltate i sindaci delle grandi città italiane. La riforma andrà a colpire persone che in Italia lavorano con contratti regolari e creerà un esercito di irregolari che non potranno essere allontanati in mancanza di accordi con i Paesi dai quali provengono e che andranno ad alimentare il mercato del lavoro nero. Cancellare la convertibilità dei permessi ottenuti in relazione alla tutela della vita privata e familiare è una delle norme più odiose, palesemente in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali: l'abbiamo ricordato

Stiamo facendo una legislazione contro i diritti e le leggi internazionali. I numeri ve li hanno riportati. La gran parte delle persone che chiede la protezione speciale, e che l'ha ottenuta, neanche arriva dagli sbarchi. Facciamo uno sforzo, fermatevi. Rinforziamo l'unitarietà del sistema di accoglienza italiano. Il Sistema accoglienza integrazione (SAI) rimanga accessibile ai richiedenti protezione e ai rifugiati; vengano ripristinati i criteri di riparto per il piano nazionale di accoglienza.

proposta. *Idem* per il presidente del Partito Popolare Europeo Weber, il quale ha dichiarato che l'Italia va aiutata, perché la situazione è assolutamente intollerabile. In questo quadro, tra Mattarella, Weber,

verso quello che, a nostro avviso, può essere un tentativo di lenire i problemi che l'immigrazione provoca quotidianamente anche alla nostra Nazione. Il piano Mattei non è qualcosa di immaginario e indefinito, ma semplicemente la constatazione che che la soluzione non può essere quella di spostare l'Africa in Europa. *(Applausi)*. Probabilmente, la cosa più giusta è eliminare alcuni europei dall'Africa, che hanno speculato con logiche postcoloniali,

sta dicendo il contrario, ma ha bisogno di coloro che riusciamo a integrare realmente; e per integrarli realmente serve poter dare loro un lavoro. Da questo punto di vista, il decreto-legge in esame inizia a compiere una vera rivoluzione, perché pone al centro della determinazione delle quote di flussi regolari dei migranti il Ministero del lavoro, cosa che non avveniva precedentemente. È questo l'orizzonte che dobbiamo assolutamente darci, anche perché, se così non fosse, chiaramente continueremmo a rifocillare la manovalanza della criminalità organizzata, come avviene per coloro che non riescono a integrarsi. D'altronde, basti pensare che abbiamo un cittadino straniero su dieci e che le nostre carceri sono, per

che seguivano l'istanza umanitaria o se fossero quelli diventati ricchi e milionari speculando sul *business* dell'immigrazione, come per troppo tempo è avvenuto in Italia.

Ciò vuol dire che un immigrato irregolare in Italia, nel momento in cui dimostra l'esistenza di rapporti sociali (ma quindi che cosa: l'iscrizione a una bocciofila, ad un sindacato o a una polisportiva), ha il diritto di non essere espulso? È chiaro che questa previsione non poteva e non può funzionare ed il decreto va esattamente in tale direzione.

difendere. Al netto dei flussi regolari, dobbiamo difendere la nostra identità, le nostre radici ellenico-romano-cristiane quello che ci hanno insegnato, appunto, gli antichi filosofi greci: l'amore per la democrazia e per il diritto; il rispetto delle minoranze, coniugato col dovere della maggioranza di prendere decisioni; il sistema giuridico romano, che ancora oggi è l'architrave del nostro diritto civile e dei nostri istituti principali; e la cultura cristiana, non nel senso confessionale o religioso,

di mettere in fila le soluzioni per un problema drammatico, che evidentemente non si può sviluppare e declinare solo sul piano nazionale, ma ha bisogno, ovviamente, anche di soluzioni continentali. E, guarda caso, da quando questo Governo è in essere, dall'Europa iniziano ad arrivare le prime risposte. Prima, invece, ogni volta che veniva sollevato il problema dell'immigrazione, l'Europa non diceva nulla. Oggi, invece, le dichiarazioni di Weber e gli atti del Parlamento europeo vanno finalmente nella direzione opposta. È quindi chiaro che, con convinzione, nonostante il vostro legittimo ostruzionismo con gli emendamenti e nonostante le vostre

sono finalmente un progetto complessivo e un comportamento corretto e responsabile, che parte dai diritti delle persone. Il primo diritto - come appunto diceva il collega prima di me - è quello di non essere costretti a emigrare - come sottolineava anche il Presidente del Consiglio qui in quest'Aula prima ancora di quello a emigrare. Nella storia in verità non è mai stato il pane ad andare verso i poveri, ma sono i poveri ad andare dove c'è il pane. Eppure, c'è uno sforzo di portare competenze e risorse in quei Paesi, di dare avvio a un piano Mattei per l'Africa, garantendo a quelle Nazioni la maggior parte degli introiti della produzione di energia; un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e Nazioni africane, che recupera allo stesso tempo il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo. Lo dimostrano i recenti viaggi in Algeria e in Etiopia del nostro Presidente del Consiglio e in Tunisia del nostro ministro degli esteri Tajani. In Giappone c'è sulla politica dei migranti. Lo dimostra l'insistenza con l'Europa per affrontare in modo unitario e strategico un tema così importante, riguardo al quale l'Italia non può certamente essere lasciata da sola; una richiesta di coinvolgimento attivo dell'Europa che sta finalmente ottenendo la dovuta attenzione e di cui noi di Forza Italia siamo stati i primi fautori. Inoltre, il Governo Meloni, Meloni, con questo decreto, incrementa i flussi regolari in entrata come mai era successo negli ultimi anni. Aumentano i rapporti di collaborazione con gli Stati di provenienza e di transito dei migranti; si colpiscono i trafficanti di uomini per ridurre i naufragi e le tragedie in mare, nonché le tante morti di persone e di bambini quello che è successo a Cutro). Lo stato d'emergenza adottato consentirà poi a tutte le strutture dello Stato di velocizzare l'*iter* di alcune procedure necessarie per avere a disposizione gli strumenti indispensabili a garantire sempre e in modo strutturale (quindi più umano e solidale) la prima accoglienza, così come ha spiegato molto bene in Commissione il sottosegretario Molteni, che ringrazio e al quale faccio i complimenti per la competenza. Mi fanno sorridere coloro i quali gridano allo scandalo per l'adozione dello strumento dell'emergenza. Sarebbe anche giusto parlare di uno strumento inappropriato per una politica che è ormai conosciuta, se non fosse che in Italia ormai tutto dev'essere affrontato con gli strumenti dell'emergenza. Figuriamoci la questione dei migranti, che arrivano oggi a decine di migliaia sulle nostre coste, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Dopo decenni di politiche di "complicazione", frutto della cultura del sospetto propria della sinistra, non riusciamo più a realizzare un'opera pubblica; non riusciamo a spendere le risorse del PNRR; non riusciamo neanche ad assumere tecnici e dipendenti nella pubblica amministrazione - e sono necessari - senza ricorrere a commissari e a norme straordinarie, che ormai stiamo recependo come ordinarie nel nostro ordinamento.

I confini non sono solo muri, a volte invalicabili, senza pietre, ma neanche linee prive di significato: racchiudono idealmente un popolo, che poi è una comunità in continua evoluzione, con valori, culture e tradizioni comuni, che si dà delle regole. Il nostro è un Paese straordinario, con un patrimonio di città storiche bellissime. Siamo eredi, forse un po' indegni, del mondo classico. I tratti caratteristici degli italiani sono proprio quelli di un'affinità elettiva con la cultura artistica la raffinatezza dei comportamenti e del pensiero, il carattere passionale e l'inclinazione verso il bello. Siamo più accoglienti e aperti rispetto agli altri. Siamo stati un popolo di navigatori e di mercanti, incline agli scambi commerciali e sociali. Sappiamo trasmettere calore umano ed è quello che ci dicono i turisti che vengono in Italia. C'è un mito nel mondo, quello degli italiani brava gente: un insieme di giovialità e di naturale inclinazione alla socialità. Nella nostra identità è insito il tratto distintivo e positivo dello spirito dell'accoglienza, che non dobbiamo perdere. Nelle nostre città ci dev'essere un posto per chi arriva da noi: non un posto qualunque chi arriva dalle miserie e dalla guerra, ma un posto d'onore, in modo che chi arriva si riconosca nei nostri valori e si senta, nello stesso tempo, a casa; quindi un posto d'onore, ma anche un posto che lo faccia sentire a casa. Sono proprio questi i temi dell'inclusione e dell'integrazione sui quali è necessario fare cospicui investimenti, se si ha a cuore la crescita sociale ed economica del nostro Paese. Siamo cittadini del presente, con alle spalle un passato che più di altri popoli europei è il risultato di migrazioni e di incroci di tante genti e culture, grazie alla posizione geografica, alla conformazione fisica del nostro Paese e al continuo movimento di popolazioni in entrata e in uscita. Io stesso provengo da una Regione, la Calabria, il cui territorio è stato abitato da una serie vastissima di popoli, quali bruzi, greci, romani, bizantini, normanni, angioini e aragonesi, solo per citarne alcuni. Davanti abbiamo un futuro, che sta in questa solida identità, ma anche nella capacità di integrare il nuovo, non solo di contenerlo spazialmente dentro i confini. Un Paese chiuso è un Paese morto. non solo un affare di buon cuore e di buon sentimento, ma anche un'esigenza di produzione di ricchezza materiale e ideale, che è utile alle nostre imprese e alla società più in generale. La sfida è riuscire a creare le condizioni per costruire una possibilità d'integrazione effettiva tra cittadini antichi e nuovi, con una prospettiva di radicamento, in modo che tutti si sentano a casa. Il nostro Paese e le nostre città vanno visti come una sorta di opera collettiva, che si rinnova continuamente, secondo una cultura di produttivo tra tradizione e innovazione. Abbiamo già assistito nella storia a questi processi. Ricordo le invasioni barbariche, che all'epoca si chiamavano migrazioni e i barbari erano i popoli che provenivano dall'Europa settentrionale, sullo sfondo della decadenza dell'Impero romano. Quando i goti avanzavano con Alarico e saccheggiavano Roma, ci fu l'azione di un santo, sant'Agostino d'Ippona, che suggerì che l'unico modo di preservare l'identità e le radici cristiane era quello di conquistare quei popoli con la cultura, come poi avvenne. Tutto questo non vuol dire assecondare la filosofia *no border*, cioè l'apertura indiscriminata dei confini, perché vanificherebbe in un colpo le idee che sono alla base di quel processo di inclusione sociale che mi è tanto caro. Neanche nella narrazione biblica

in entrata e per andare incontro alle richieste dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e a quelle di Confindustria, per assicurare alle imprese i lavoratori e per

in questo edificio, durante una riunione di Gruppo che i colleghi ricorderanno, propose addirittura di mettere a disposizione le case sfitte per le persone che arrivavano nelle

ho preferito non sottoscrivere l'emendamento che riguarda la protezione speciale: pur essendo sicuro dei buoni intenti e della buona fede di chi lo propone, volta a ridurre i pretesti per l'immigrazione clandestina, avevo e ho dubbi riguardo ad alcuni effetti che potrebbero generarsi nei confronti di chi è già integrato, di chi lavora e ha creato una famiglia nel nostro Paese. Abbiamo letto sui giornali alcune storie che mi hanno fatto anche riflettere rispetto a questo. Purtroppo non è stato possibile un confronto sereno con l'opposizione, perché in 1a Commissione sono stati presentati, in modo strumentale e pretestuoso, circa 400 emendamenti, che hanno creato un teatrino, per esigenze di propaganda elettorale e di fatto hanno impedito la discussione nel merito rispetto a questo punto così importante. Nonostante il presidente Balboni abbia guidato quella Commissione, non siamo riusciti poi a sviluppare questi argomenti. Affido quindi queste mie riflessioni al Governo e al presidente del Consiglio Meloni, nella consapevolezza che sapranno tenerle nel giusto conto e, nel caso di possibili distorsioni, correggere con il buonsenso e l'umanità che li contraddistinguono le problematicità che potrebbero verificarsi. Nonostante le buone intenzioni e il buon lavoro svolto dal Governo, nessuno in questo caso può dire di avere una ricetta perfetta per la soluzione di un problema epocale così complesso.

ricorderanno, che generò polemiche. Anche in quel caso, come oggi, l'Italia non fece un passo indietro sul fronte dell'accoglienza. Allora come oggi, l'Italia fu costretta a urlare all'intera Europa a squarciagola, è vero che la lotta all'immigrazione è un principio di legalità e di sicurezza continentale, ma che non può essere solamente una battaglia di facciata.

"pattugliamento" - pensate un po' - attuò un vero e proprio blocco navale, che portò anche a una tragedia: era il marzo del 1997, un venerdì santo per essere esatti, quando, a seguito di una collisione tra un'imbarcazione carica di migranti e un nostro mezzo di pattugliamento, morirono 81 persone.

esso non aveva, com'è stato ampiamente dimostrato (anzi, è stato fatto tutto il possibile per salvare vite umane). Il buonismo di facciata al quale abbiamo assistito in questi anni non ha risolto i problemi non ha evitato le morti in mare, né le nefaste conseguenze dell'immigrazione irregolare, che nei grandi centri urbani, nelle stazioni e nelle periferie si è trasformata in una bomba sociale che pagano i cittadini in termini di sicurezza, serenità e vivibilità. Chi ha propugnato le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati a tutti i costi non si è curato delle conseguenze dell'immigrazione irregolare, né del destino di migliaia di stranieri che, senza casa, senza lavoro, senza documenti e senza dignità, hanno visto il sogno italiano e - mi consenta - europeo diventare un incubo per la sopravvivenza. E, quando devi sopravvivere, Presidente, il pericolo di sconfinare nell'illegalità e nel crimine è a un passo, come purtroppo è accaduto e accadrà. e qui mi vergogno - ha anche speculato sull'accoglienza, ha ingrassato le cooperative e ha intercettato finanziamenti pubblici, allargando non il cuore per accogliere, formare e integrare, ma il portafogli per drenare contributi alla faccia dell'umanità e dei buoni sentimenti. *(Applausi)*. Il caso che ha coinvolto la famiglia del collega Soumahoro è emblematico. Sono un garantista sia per indole sia per professione,

Sin qui le politiche dei porti aperti e degli ingressi indiscriminati hanno fallito. Occorre rovesciare la prospettiva, devono esistere un diritto a non emigrare, ma anche la possibilità per un cittadino del Continente africano di scegliere di rimanere nella propria terra e di avere un lavoro e una crescita economica. Il piano Mattei per l'Africa è la *summa* di tutto ciò: tutto ciò: vuol dire cooperazione, scambi commerciali e collaborazione economica, politica e sociale per tanti Paesi ricchi di risorse e di forza lavoro, che può trovare sbocco proprio in Africa, promuovendo quindi sviluppo e migliori condizioni di vita e crescita. Il piano Mattei guarda al Mediterraneo con una prospettiva nuova, per certi versi obbligata. Il dominio cinese sull'Africa e sulle sue materie prime è un altro tema che impone una riflessione

dal primo gennaio all'11 aprile 2023 sono arrivati in Italia 31.292 migranti, con un incremento pari al 294,7 rispetto allo stesso periodo del 2022 (7.928 migranti). Se dovesse mantenersi questo *trend,* si stima che per la fine dell'anno potremmo arrivare a oltre 400.000 nuovi arrivi. L'incremento dei flussi ha dunque portato a un insostenibile sovraffollamento dei centri di prima accoglienza, in particolare presso l'*hotspot* di Lampedusa, che ha una capienza di soli 389 posti e nei giorni tra il 10 e il 12 e dal 24 al 26 marzo ha registrato presenze fino a 3.000 persone. Ad oggi, il totale delle persone in accoglienza in Italia è pari a 114.643 migranti. Pensate veramente, colleghi dell'opposizione, che davanti a questi numeri basti aprire le braccia e sorridere per governare un cataclisma come questo? Basta semplicemente dire di venire in Italia sorridendo, per poter dare la percezione che qui c'è spazio per tutti? Ho letto e ascoltato tante polemiche sulla protezione speciale. Non serve un'ulteriore via di protezione che, reintrodotta dal secondo Governo Conte, anche per calamità naturali o cure mediche rende automatico il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di due anni, ma che in un solo anno ha aumentato in maniera consistente le partenze senza generare lavoro. lavoro. Per invertire la rotta servono due tasselli: visione e programmazione. La visione è quella del piano Mattei, secondo il concetto che il primo diritto è quello di non essere costretti a emigrare. La programmazione è racchiusa in questo decreto-legge che pone un progetto chiaro: in Italia si entra, si arriva e si lavora solo in maniera regolare, passando per la procedura di legge. *(Applausi)*. Chi vuole aggirare queste procedure non sarà accolto; chi vuole delinquere facendo il trafficante di esseri umani al soldo di associazioni criminali sarà severamente punito. Questo è un messaggio chiaro che il Governo lancia alla Nazione. Grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni il tema dell'immigrazione ha acquistato una centralità europea e di questo siamo tutti consapevoli. i trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti; i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte; le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Basta morte e dolore, signor Presidente, su questo siamo tutti d'accordo, ma basta anche nascondersi dietro un falso buonismo. Affrontiamo da Nazione seria quale siamo un tema complesso, con una visione di lunga gittata, anche per la dignità di chi arriva in Italia e ha il diritto di starci.

contro non solo le opposizioni, ma anche le associazioni, le ONG, i sindacati e addirittura Magistratura democratica, che ieri ha aderito alla manifestazione; e poi ovviamente tutti i sindaci del PD,

della sinistra che, tra le critiche più dure che abbiamo sentito, ci taccia di non avere umanità, di essere cinici. Più volte anche in quest'Aula siamo stati invitati a guardare negli occhi i migranti che sbarcano, come se fossimo del tutto insensibili e disinteressati alle loro vite e al loro destino. destino. Credo invece che gli unici davvero disinteressati alle vite e al destino della povera gente che sbarca in Italia siate proprio voi, voi, con il vostro buonismo di facciata, messo sempre in bella mostra davanti a microfono e telecamere ogni qualvolta si registra una tragedia come quella di Cutro,

Innanzi tutto, tra le 15 rotte attuali, quella del Mediterraneo è la più pericolosa. E non siamo noi a dirlo, ma dell'ONU: dal 2014 ad oggi, quasi la metà dei migranti morti o dispersi nel mondo si è registrata nel solo nostro mare, oltre 27.000 persone; nel 2022 il numero dei dispersi ha superato il numero dei morti accertati, doppiandolo, e nei soli primi tre mesi del 2023 abbiamo registrato, con una stima al ribasso, oltre 500 persone annegate. Di fronte a questi numeri, solo chi non vuol vedere in faccia la realtà può permettersi il lusso di tacciarci di disumanità e insensibilità. Come pensate di porre rimedio alla pericolosità di questa rotta e impedire le morti in mare? Solo con i soccorsi, spesso proibitivi e a volte impossibili per tutti, nonostante il lavoro incessante della Guardia di finanza e di altre Forze dell'ordine, che voglio qui ringraziare, a nome del mio Gruppo? Pensate forse che, com'è stato lasciato solo dall'Europa, nonostante i continui appelli, l'ultimo dei quali del presidente Mattarella, che voglio ringraziare per la netta posizione espressa in Polonia, possa davvero avere la forza d'intercettare e intervenire su ogni partenza per soccorrere tutti i migranti che si imbarcano e poi assisterli anche a terra? Io vengo da una delle Regioni di maggior approdo, la Calabria, e conosco da vicino l'abnegazione e l'impegno senza sosta di agenti e militari, che al lavoro della macchina dei soccorsi sommano anche il lavoro ordinario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Pensate che si possa continuare a far pesare il carico di salvataggio e assistenza su quelle stesse risorse, che sono insufficienti ancora oggi a coprire le esigenze del territorio, nonostante il potenziamento degli organici che noi abbiamo disposto disposto come Lega e come centrodestra? Ma voi cos'avete fatto finora, se non parole? Dimostrate sempre - è vero - una grande sollecitudine nel preoccuparvi, ma solo del primo momento dell'immigrazione, cioè i viaggi dei disperati, usarli contro gli avversari politici, salvo poi dimenticarvene in un momento successivo, quello dell'accoglienza. Il senatore Parrini avrebbe dovuto vergognarsi in passato, non certo oggi. Le vostre parole oggi sono più vuote e piene di ipocrisia e a dimostrarlo sono sono certamente altri dati, quelli sugli sbarchi e sui morti negli anni passati. L'unico momento in cui li abbiamo drasticamente ridotti e il numero dei morti in mare è stato il più basso di tutti gli anni e di sempre è stato quando a ricoprire la carica di Ministro dell'interno era il senatore Matteo Salvini *(Applausi)*. È un fatto incontrovertibile, non propaganda elettorale, com'è stato anche detto in quest'Aula. È la riprova che frenare le partenze significa salvare vite umane: ecco perché le vostre accuse s'infrangono, come onde del mare, proprio contro la verità dei numeri. Le nostre politiche di allora, come quelle di oggi, servono non a salvare noi italiani, ma loro, i migranti, da viaggi che si rivelano (non sappiamo nemmeno quanto) e da una vita misera o comunque disperata, perché migliaia di persone arrivano qui pensando di trovare la loro America e trovano invece fame, disoccupazione ed emarginazione, dato che il sistema non riesce ad assorbirle e integrarle tutte, regalando loro un'esistenza dignitosa come avrebbero diritto. Allora, a cosa puntiamo con questo decreto-legge? Non vogliamo certo bloccare le migrazioni, caro senatore Lombardo. Sappiamo bene della necessità dei flussi migratori sul nostro territorio. Saremmo sciocchi anche solo a pensarlo e non sarebbe neppure etico, oltre che contrario a un mondo sempre più globalizzato. Quello che intendiamo fare oggi è gestire le migrazioni, cosa che non avete mai fatto. Noi vogliamo accompagnarle, governarle e soprattutto regolarizzarle, perché solo così possiamo evitare i morti in mare, ma soprattutto offrire a tutti coloro che riusciamo ad accogliere. È appunto in questa direzione che vanno le norme che siamo qui a discutere e i nostri emendamenti, tutti volti - da un lato - a contrastare l'immigrazione irregolare, in modo anche indiretto, e quindi sottraendo ai trafficanti di uomini la merce che serve loro solo per lucrare soldi, e - dall'altro - a semplificare e velocizzare le procedure per l'immigrazione regolare, così da garantire a chi arriva una vera opportunità di riscatto. Per farlo bisogna chiaramente partire da un contingentamento degli ingressi: prevediamo quote preferenziali per chi proviene da Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi dei traffici irregolari; e rendere edotti di questi rischi coloro che scappano dal proprio Paese significa prevenire la possibilità di farli cadere nelle mani dei trafficanti. Cosa c'è di sbagliato in una norma che aiuta i migranti a cercare canali leciti per partire in cerca di futuro? Ancora una volta, con questo decreto-legge, il Governo dimostra una grandissima capacità di vedere oltre; dimostra vero interesse e la voglia di dare davvero l'occasione di una vita migliore a chi trasmigra, evitandogli come unico sbocco la strada o l'arruolamento nelle fila della criminalità. È vero che un detenuto su tre nelle carceri è straniero, ma, senatrice Maiorino, non è certo per colpa nostra oggi. In tema di lavoro agricolo - che ovviamente assorbe tanti migranti - il Governo, snellendo le procedure, da un lato, tutela la forza lavoro, cioè i migranti stessi, e, dall'altro

quando, come primo atto, ho avviato un progetto - ancora in corso - di smantellamento della tristemente nota baraccopoli di San Ferdinando per sostituirla con un villaggio ecosolidale, con tutti i crismi, a sostegno dei braccianti. Di questo nessuno in quindici anni si è mai occupato,

d'emergenza, il nostro ministro Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni, che ringrazio per l'impegno profuso. Voi cos'avete fatto invece finora, nelle vostre Regioni rosse come la Puglia, se non riempirvi la bocca

non solo delle morti in mare, ma anche del degrado in cui la maggior parte dei migranti si trova a vivere oggi per l'impossibilità di offrire a tutti un'esistenza dignitosa. Sono anzi le maglie larghissime che tanto amate, a volte, a incattivire questa povera gente che, una volta sul nostro territorio, finisce rinchiusa senza prospettive in centri di accoglienza o di permanenza sovraffollati e ingestibili, senza dignità e men che meno libertà. Siete voi a consegnarli a questa vita miserabile; ancora voi a considerarli numeri e non persone. Grazie a noi, invece, lo Stato oggi diventa finalmente protagonista e soggetto attivo, che vuole guidare attivamente il percorso dei migranti, anziché subire passivamente il loro arrivo e l'azione criminale dei trafficanti. Voi parlate, noi agiamo nell'interesse reale di tutti: questa è la differenza.

Tutti noi, ancora oggi, ricordiamo quella tragedia, che ha un po' graffiato e scalfito i nostri cuori e la nostra sensibilità, che ha segnato profondamente la vita di donne e uomini che si sono visti restituire dal mare i corpi inermi e senza vita di altri esseri umani.

la profonda tristezza negli occhi di chi ha vissuto quegli attimi di inumanità; le immagini dei giocattoli dei bambini che hanno perso la vita in mare; gli occhi smarriti dei bambini che avevano perso i genitori e di genitori che avevano perso i figli. Ho parlato con quelle persone, è per questo che la discussione che stiamo facendo mi sembra veramente surreale. Pensare che quella conferenza e che questo provvedimento siano stati la risposta che il Governo ha inteso dare a quella tragedia rende chiare ancor di più la confusione e l'assoluta strumentalità della maggioranza. In Commissione non siete riusciti a sciogliere i vostri nodi e il provvedimento è arrivato in Aula senza relatore. Prima di chiedere risposta ai nodi che attanagliano la maggioranza, faccio però l'ennesimo appello che è arrivato non solo dai banchi dell'opposizione, ma anche dal Paese, da quelli che ieri l'hanno chiesto, non da quelli che fanno i soldi, ma da quelli che aprono il loro cuore all'accoglienza vera. Certo, quando non ci sono accoglienze vere, è giusto che ci siano indagini e che si chieda la verità, ma la maggioranza di quelle associazioni ci ha chiesto di essere ascoltata. Su quella tragedia non abbiamo ancora saputo la verità. Non vogliamo diventare il Paese che rimanda sempre la ricerca della verità fino a farla entrare nell'oblio, il lungo tempo che ci deve far dimenticare. Oggi, a gran voce, chiediamo ancora una volta al Governo che venga fatta chiarezza, perché sono morte più di 100 persone (i cadaveri recuperati sono 94). Il Governo non è ancora stato in grado di spiegare per quale ragione non si sono attivati i soccorsi. Vogliamo solo saperlo. Mentre il mare restituiva i cadaveri, voi organizzavate una conferenza stampa: l'ennesimo teatrino, l'ennesima occasione per usare l'immigrazione come tema di propaganda elettorale. Eccolo qui il risultato, è davanti ai nostri occhi: in nome della propaganda, fate a gara con chi la spara più grossa. Sentiamo parlare di allarme, leggo di Ministri della Repubblica che parlano di sostituzione etnica. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Le parole hanno una responsabilità e un Ministro che parla

è nato mentre il mare ci restituiva cadaveri di donne, uomini e bambini: esseri umani che scappavano dalla disperazione e che non avevano alcuna intenzione di partecipare a fantomatiche sostituzioni etniche. Un riferimento particolare poi voglio fare a proposito dell'eliminazione della cosiddetta protezione speciale. Tanti altri colleghi si sono soffermati sul punto. Per il presidente Meloni il nostro Paese offrirebbe una protezione ulteriore rispetto a ciò che accade nel resto d'Europa. A suo avviso, un fatto ingiusto; a nostro avviso, una falsità colossale, ma lo avete detto anche voi, cari colleghi senatori. Vi invito a leggere - oppure a rileggere, per chi lo ha già fatto e magari lo ha dimenticato - il *dossier* Senato compilato nel 2018 in occasione della conversione in legge dei decreti Salvini, che spiega in maniera abbastanza semplice e chiara la lunga lista di protezioni complementari presenti presenti in 18 Paesi, oltre a quella dell'asilo politico e della protezione sussidiaria. In Europa, 18 Paesi su 27 hanno forme di protezione umanitaria analoghe alle nostre. Allora, delle due l'una: o il presidente Meloni è in malafede oppure non conosce di ciò di cui parla. In entrambi i casi, siamo di fronte a un fatto grave, perché dovremmo smetterla di usare l'immigrazione come terreno di una becera propaganda politica. Si tratta di esseri umani che scappano della guerra, dalla povertà e dalla fame e hanno il diritto di sognare una vita migliore.

su dieci dei permessi totali rilasciati, che viaggiano perfettamente in linea con la media europea, intorno al 40 per cento rispetto alle richieste. La Germania, che riconosce forme di protezione umanitaria molto simili alle nostre, nel 2022 ha concesso più di 30.000 protezioni complementari, circa il 25 per cento del totale dei permessi rilasciati. La Spagna, Paese non proprio celebre per la facile concessione dei permessi, nel 2022 conta più di 20.000 il doppio dell'Italia, più della metà dei permessi di soggiorno concessi. Persino l'Olanda, l'Austria, l'Ungheria e la Grecia, ossia Paesi solitamente ostili a politiche di solidarietà, prevedono forme di protezione umanitaria. Allora, signor Presidente, diciamo la verità: siamo di fronte all'ennesima pantomima, a un provvedimento palesemente incostituzionale, che permette alle forze politiche che compongono la maggioranza di sfuggire alle vere questioni su cui i cittadini aspettano risposte. Servono soluzioni concrete per una vera politica d'integrazione e gestione dei flussi migratori e in questo decreto non le vediamo. Attendiamo risposte sull'attuazione del PNRR, sul sostegno alla povertà, sulle politiche di sostegno alla natalità, sulla lotta al cambiamento climatico, sulle riforme e sul contrasto alla criminalità organizzata e approfitto qui per ricordare che la Commissione antimafia non è stata ancora convocata, mentre credo che ce ne sarebbe un gran bisogno. Ecco, di fronte alle mancanza del Governo, la maggioranza si rifugia nel suo cavallo di battaglia, la propaganda populista sull'immigrazione. La verità, però, è che con questo provvedimento non fate altro che alimentare un clima di odio e paura; una paura che stravolge improvvisamente la vita degli oltre 10.000 stranieri che lo scorso anno hanno ottenuto il permesso umanitario in virtù della protezione speciale assicurata a chi è vittima di persecuzione e torture, per motivi di salute a chi si sente abbandonato. Abbandonare persone fragili e sofferenti, tuttavia, è uno dei peggiori crimini che un essere umano possa commettere. Fermatevi. Non c'è nulla di logico, né di umano: state solo peggiorando la situazione degli uffici giudiziari, che saranno chiamati a dirimere i ricorsi. State solo rubando il futuro a migliaia di persone; state solo creando un esercito di invisibili senza protezione e senza diritti, e di irregolari decretati per legge, pronti a essere manovalanza per la criminalità organizzata. Sulla pelle di queste persone si sta giocando una partita di civiltà, ma voi avete deciso di non scendere in campo. Insomma, prendetevi un attimo ripensate alla ragione per la quale questo decreto si chiama Cutro. Ripensiamo allora a quei cadaveri, ripensate alle storie di chi oggi aggiungerà ulteriori difficoltà alle proprie sofferenze. Fatelo e può darsi che vi ricorderete di avere occhi giusti e cuore aperto per ritornare a essere umani. *(Applausi)*.

alcune prese di posizione che appaiono più che strumentali. Anche nell'ultimo intervento si è parlato della strumentalizzazione che il centrodestra, Fratelli d'Italia e il Governo avrebbero fatto sulla tragedia di Cutro. Cutro. Vi invito però - se ve lo siete già dimenticati - ad andare a rileggere quello che dichiaravate in quei giorni su Cutro, quello che avete cercato di portare come strumentalizzazione di una tragedia assoluta vista nei nostri mari, i tentativi di accusare questo e quello, finanche la Guardia costiera per quello che era accaduto. Allora, se non vogliamo parlare di strumentalizzazione e di immigrazione solo per fini per fini di propaganda, anche non esclusivamente elettorale, ma per risolvere il problema, ciascuno con le proprie idee e con le proprie diversità, forse prima di accusare gli altri bisognerebbe farsi un esame di coscienza su chi è stato il primo a

una grande dissimulazione in questi giorni e c'è oggi in Aula, nel tentativo di far credere che con questo decreto si voglia eliminare la protezione speciale, anche se non si elimina rispetto a quelli che ci sono in tutto il resto d'Europa. La chiamiamo protezione umanitaria, come sarebbe corretto fare. E sappiamo benissimo - forse più noi che voi, visto che ne continuate a parlare in termini negativi - che tra

quella che voi definite speciale e che noi definiamo oggi umanitaria, è lasciata alla discrezionalità degli Stati. Non vi sto ad elencare quello che negli altri Stati europei è previsto per la protezione umanitaria, ma vi dico che con questo decreto-legge l'Italia si porta a un livello superiore a quello degli altri Stati europei. Sapete qual è la grande differenza? Che saranno tassativamente elencati i motivi per cui la protezione umanitaria potrà essere concessa.

Di queste, è vero che solo 10.800 circa hanno avuto la protezione speciale umanitaria, circa 7.000 hanno avuto la protezione sussidiaria e 6.100 lo *status* di rifugiati. Rimangono, nel solo 2022, 83.000 persone che non sappiamo dove siano finite, che non hanno nessun titolo a rimanere sul nostro territorio e che, sommate alle centinaia di migliaia di persone degli anni precedenti, formano

nei campi a cui faceva riferimento prima l'esponente della Lega e che voi forse, quando governavate, avete finto che non esistessero; campi in cui non è neanche lontanamente possibile individuare decine di migliaia di persone ammassate senza alcuna possibilità di sussistenza che non sia lavoro nero e sfruttamento; migliaia di persone che vivono attorno alle stazioni delle grandi città, a Roma, a Milano e da altre parti,

Stati. Quando sostenete di aumentare l'immigrazione dando diritti a tutti, vi chiedo: quali sono i diritti a cui pensate? Il diritto di vivere in una baracca, senza acqua potabile, senza fognature, senza cibo e senza fuoco? Sono questi i diritti a cui avete pensato negli ultimi dieci anni in cui siete stati al Governo? Sento parlare di immigrazione di massa, ma a cosa serve l'immigrazione di massa, se non ci sono né le risorse, né i modi per governarla? Forse a ingrossare ma forse anche a ingrassare - le cooperative che per anni hanno mangiato sull'immigrazione? Mi dico allora che questo decreto-legge è un forte passo avanti,

per l'Italia nella ricerca della *governance* dell'immigrazione, ma anche per dare a chi viene in Italia quella dignità di donna, di uomo e di bambino che dovrebbero avere tutte le persone che scelgono il nostro Paese per vivere.

al lavoro queste persone che nascono ci andranno fra diciott'anni. Nel frattempo, abbiamo imprese che richiedono più di 200.000 immigrati per svolgere lavori quest'estate e quest'anno. E noi cosa gli rispondiamo? Questo non lo dico io. In agricoltura ci sarebbe bisogno di 100.000 lavoratori, che non si trovano. Nell'agroturismo, la Confesercenti riferisce di un buco di 50.000 lavoratori. Ancora,

rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, è già stato detto molto dal mio collega di partito e di Gruppo Marco Lombardo nei suoi interventi precedenti. del Governo, dovreste davvero cambiare nome a questo decreto. È un decreto sicurezza-*ter*, come più volte è stato detto nei tanti interventi che ci sono stati da parte dei colleghi. Prima di tutto, per il rispetto che si deve alle persone che non ci sono più e che sono morte nella tragedia di Cutro e ai bambini di cui poi nei giorni successivi abbiamo visto le

concreti e razionali, guardare veramente la fotografia che abbiamo oggi del Paese, ma non solo del paese Italia, bensì dell'Europa. Le parole sono importanti. Quando un importante Ministro del Governo parla di sostituzione etnica - e anche qui, tra i banchi della maggioranza, abbiamo ancora

allo spirito di umanità, di solidarietà e di accoglienza che appartiene, questo sì, all'identità stessa del paese Italia. Volete tornare ai decreti Salvini? Ditelo apertamente. Volete tornare a quelle norme che assolutamente hanno cancellato i diritti fondamentali e le libertà individuali delle persone, senza portare a nessun risultato rispetto alla questione degli sbarchi? Questa è la verità. finitela di essere in campagna elettorale in modo permanente, perché la campagna elettorale è finita e i problemi rimangono tutti tali e quali. Non c'è un tema di emergenza, come l'avete chiamata voi;

Dobbiamo parlare di temi, questi sì, prioritari, come ha ricordato prima il collega Lombardo, legati alla denatalità. Quando ci sono 400.000 bambini in meno nel nostro Paese e quando il 25 per cento della popolazione è *over* 65, allora ci dobbiamo fare delle domande. Come ricostruiamo un sistema di *welfare* equilibrato rispetto alle esigenze del nostro Paese? Come possiamo tenere assieme la richiesta delle imprese e degli imprenditori, che chiedono manodopera in tanti settori strategici del nostro Paese, che porterebbe quindi soltanto benefici e un aumento del PIL? Come possiamo tenere il tema della demografia? Sono tanti i temi su cui ci dovremmo interrogare: quali politiche sociali e quali politiche attuare per tenere assieme un sistema che già oggi non regge più come sistema di *welfare*? Purtroppo, ancora una volta, l'impostazione del Governo è sempre la stessa: si alza una bandierina e si dice che c'è un problema di allarme sociale e di emergenza, ma poi non si fa niente. Addirittura, fate una cosa ancora più grave: continuate a fare decreti-legge (decretazione d'urgenza) e poi cambiate le norme in corso d'opera, cambiate gli stessi decreti quando già sono state scritte le norme.

C'è una richiesta pazzesca: ci chiedono di non abbandonare e di non smantellare il sistema di protezione speciale. Ricordo anche che questa è una misura che ormai esiste in 18 Paesi europei su 27, praticamente in tutti i Paesi dell'Europa occidentale. Circa il 50 per cento dei migranti è costituito da nuclei familiari. Senza la protezione speciale, non solo ci sarebbe una costante lesione dei diritti individuali, ma queste persone rimarrebbero condannate ad essere invisibili. In questo quadro, semmai, occorre ripensare anche il sistema d'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che è un grande tema di cui non parlate. Ecco perché serve un piano nazionale d'accoglienza pubblico, trasparente e professionale, per consentire percorsi tutelati e dignitosi, anche per le persone richiedenti protezione internazionale. Servono procedure d'identificazione e *screening* sanitario: così si fa sicurezza sociale, non con la propaganda e con la paura dell'invasione dello straniero.

percorso d'integrazione di queste persone e di regolarizzazione di coloro che già vivono nel nostro Paese. Soprattutto, non ci possiamo isolare dal resto dell'Europa, come invece stiamo facendo. Dov'è l'autorevolezza dell'Italia?

la propaganda, guardiamo in faccia la realtà e parliamo con i nostri Comuni e con le nostre comunità; altrimenti, nessuno fermerà i flussi migratori. Di fronte al pericolo della morte, alle violenze e alle torture, cosa farebbe un cittadino normale? Cosa farebbe ognuno di noi, se si trovasse in una situazione del genere? Ecco perché bisogna essere autorevoli in Europa, cambiare gli accordi dove non vanno bene e farne con i Paesi di origine di questi cittadini e di queste persone che scappano dalle guerre, dai conflitti e dalle violenze.

Serve infatti all'Italia e a tutta l'Europa trovare non solo una dimensione umanitaria, ma ricostruire e riconsiderare un sistema di *welfare* che oggi già non regge più. Concludo, signora Presidente, non solo citando la necessità dello *screening* sanitario, come ho detto prima, la cura di familiari gravemente malati, la conclusione di formazione scolastica o professionale, l'aiuto alle vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo oppure di discriminazioni razziali o per motivi di orientamento sessuale (perché questo si fa in Germania, in Spagna, in Francia, in Olanda e persino in Austria e in Ungheria, Paese a cui siete molto legati),

Se non si mette un po' di ordine fra i vari strumenti giuridici attraverso i quali è possibile arrivare e restare legalmente in Italia, anche l'integrazione degli immigrati diventa difficile. Oltre a questo, si potenziano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che svolgono la tratta di esseri umani. Viene infatti previsto anche l'inasprimento delle pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina. Dopo la tragedia di Cutro, che ovviamente ha toccato tutti noi profondamente, rispetto al ruolo di chi traffica esseri umani è stata introdotta la nuova fattispecie di reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia d'immigrazione clandestina. Purtroppo, nonostante la buona volontà dei senatori della maggioranza in 1a Commissione e nonostante il lavoro puntuale e certosino del presidente Balboni e la presenza assidua del sottosegretario Molteni, non siamo riusciti a terminare l'esame. Sarà quindi il voto dell'Assemblea a valutare - speriamo positivamente - gli emendamenti sostenuti dalla maggioranza che puntano a migliorare ulteriormente il testo del decreto. Alcune di queste disposizioni interessano più direttamente la mia Sicilia, in particolare Lampedusa, dove sarà possibile attivare postazioni della Croce Rossa e del 118. Questo dimostra l'attenzione del Governo innanzitutto per l'accoglienza dignitosa e appropriata in un'isola martoriata da troppi anni di arrivi incondizionati. Lampedusa, Presidente, meriterebbe il premio Nobel per la pace per essersi fatta carico per oltre trent'anni di sbarchi sulle proprie coste, di misure di accoglienza assolutamente straordinarie, ma elargite con grande generosità. Va detto subito che comunque Forza Italia si è fatta carico anche di molte proposte di modifica per dare un quadro di maggiore umanità, facendo proprie le proposte di chi professionalmente si occupa di rifugiati. Avremmo valutato positivamente il confronto anche con le proposte dell'opposizione, perché questo tipo di regole è sempre bene scriverle insieme, ma purtroppo questo non è avvenuto. avvenuto. L'opposizione ha preferito chiudersi nell'ostruzionismo, senza valutare che misure per una più puntuale gestione dei flussi migratori riguardano tutti e non solo l'attuale Governo del Paese. Vorrei però tornare su quello che reputiamo uno dei punti più qualificanti del decreto: la revisione del meccanismo dei flussi per andare incontro alle esigenze delle imprese e alla richiesta di manodopera stagionale. Attraverso le nuove regole, la programmazione dei flussi di ingresso legale nel nostro Paese dei lavoratori stranieri viene realizzata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. C'è una precisa programmazione legata alle esigenze delle imprese, quindi le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato vengono definite per un intero triennio.

vengono coinvolti vari attori interessati all'arrivo della manodopera. Viene previsto il coinvolgimento del Parlamento e delle Commissioni competenti, che ovviamente potranno audire i rappresentanti delle categorie dei diversi territori per sentirne le esigenze. Si fissano poi alcuni criteri precisi che incidono anche sugli arrivi irregolari. L'ulteriore passo in avanti ora previsto è la semplificazione delle procedure per avviare il rapporto di lavoro degli stranieri con le aziende italiane. Viene introdotta un'accelerazione della procedura di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato, soprattutto per le esigenze di carattere stagionale. Sono quindi previsti gli ingressi fuori quota per gli stranieri che, nel Paese di origine, hanno superato i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia. Viene modificata anche la durata dei permessi di soggiorno, che possono durare fino a tre anni anziché due, per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. Si affronta anche il problema della protezione del mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, con disposizioni che rafforzano il ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per ottimizzare la sua azione di contrasto alle frodi, al personale impegnato viene assegnata la qualifica di ufficiale o di agenti di polizia giudiziaria. Sono state inserite disposizioni per il commissariamento della gestione dei centri per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri e comunque per farne proseguire il funzionamento. Il decreto-legge in esame, con le modifiche apportate dalla maggioranza, punta a dare maggiore certezza sia allo straniero che intende inserirsi in modo regolare nel nostro tessuto sociale, sia ai cittadini italiani che chiedono sempre garanzie di legalità e sicurezza. direi che dopo tanti *slogan* propagandistici è venuto il momento di fare i conti con la realtà la realtà che, cari amici della maggioranza, è ben diversa da quella che avete prospettato nei vostri *slogan* e nella campagna elettorale. La realtà è diversa e ci dice una cosa

di tempo non ha prodotto nessun effetto, almeno di quelli che avevate dichiarato nella vostra propaganda: non ha ridotto gli sbarchi, che addirittura sono aumentati, tanto che siete arrivati a dichiarare lo stato di emergenza.

che, ruggendo più forte degli altri animali, avrebbero avuto sempre ragione, avrebbero sempre avuto vittoria; tuttavia, i dinosauri sono proprio quelli che si sono estinti

con il rigore logico, con ponderazione, avendo anche una visione più ampia rispetto a questa visione così frettolosa, che non riesce a offrire soluzioni, perché non affronta il problema alle radici.

perché non si può affrontare un tema di così grande portata nella fretta di dare una risposta elettorale. Manca una visione programmatica. Non è una novità l'immigrazione e non sarà una novità l'aumento dei flussi migratori, che - come già sappiamo - si incrementerà nel tempo.

Ormai tutti hanno capito che la promessa di avere le soluzioni pronte in tasca, quelle che sbandieravate in campagna elettorale, in realtà è un nulla di fatto, sono parole al vento; neppure il ruggito di un dinosauro, semmai è un cagnolino che sta abbaiando di fronte al silenzio di una pantera, diciamoci la verità. Vedete, anche questa dichiarazione di emergenza, se manca una visione programmatica, assomiglia un po' troppo a una dichiarazione di sconfitta, perché non avete offerto alcun tipo di soluzione credibile al problema. Presidente, mi lasci fare un'osservazione: francamente non ci fidiamo molto di affidare la gestione di un'emergenza a una forza di maggioranza che - vorrei ricordarlo - nella scorsa legislatura non sapeva neanche cosa fosse un'emergenza. Dai banchi dell'opposizione l'attuale maggioranza ci accusava e accusava il Governo Conte di aver inventato un virus che non esisteva, il Covid. Dicevano che non dovevamo dichiarare lo stato d'emergenza e - pensate - lo dicevano in un momento in cui il sistema sanitario nazionale era al collasso: non avevamo i vaccini, né le mascherine e dovevamo difenderci. In quel momento, qual era la soluzione offerta da chi oggi è nella maggioranza? Non fare nulla, dimenticarcelo. Immaginate in che situazione ci saremmo trovati oggi, se non fosse stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Si può utilizzare, è una scorciatoia legislativa, ma su un tema così delicato, su cui l'opinione pubblica è divisa, vogliamo darci il tempo per una maggiore ponderazione? Vogliamo consentire anche ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento di emendare, se hanno qualche idea importante da mettere in campo? Al di là di questo provvedimento, quello che mi preoccupa è l'insieme delle politiche migratorie che la maggioranza vuole mettere in campo, perché non servono a nulla. Si fa un intervento sulle ONG e ci si preoccupa che si possa fare un doppio salvataggio in mare. Che sarà mai? Si fa un decreto flussi, ci si rende conto che poi, tutto sommato, alle imprese servono i migranti e si consente l'ingresso di 80.000 migranti regolari, ma non si fa nulla per la cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre. terre. Se si vuole fare cooperazione internazionale, bisogna cercare di creare le condizioni minime per la sopravvivenza. Qui c'è un problema: mancano gli ospedali e le scuole, la gente fugge anche per ragioni di salute e dalle guerre.

Vorrei entrare nel merito del provvedimento, perché davvero, se non ha avuto effetti materiali o non ha avuto quelli che sperava il Governo, di effetti devastanti sul sistema giudiziario ne ha avuti anche troppi. Partiamo da un elemento che è emerso: come ha detto prima una collega della maggioranza, c'è stato l'inasprimento delle pene. Benissimo, voi sapete che abbiamo un ordinamento giuridico che è nato sulla base di un equilibrio sanzionatorio: a fronte di un fatto più grave dell'altro, il fatto più grave deve avere una sanzione maggiore, com'è ovvio. com'è ovvio. Colleghi, fate attenzione a questo, ve lo dico da giurista, non da politico: non si può prevedere la sanzione della reclusione, con un massimo edittale di trent'anni, per un reato colposo. *(Applausi)*. Cosa facciamo per i reati volontari?

si chiama dolo - un conto è la colpa, che è negligenza, imprudenza, imperizia, e un altro conto è la preterintenzione. Non possiamo stravolgere quell'equilibrio che esiste da quando fu creato addirittura il codice Rocco. Così facendo, si fa soltanto la voce grossa, che non è quella del dinosauro, ma quella di un cagnolino. Altro punto: volete inasprire le pene? Benissimo, è legittimo farlo, ma siamo in un ordinamento giuridico in cui si rispetta anche la Costituzione. Mi sono preoccupato, ad esempio, quando ho visto le sanzioni. Per carità, potete metterle, ma, come sapete, devono avere una funzione retributiva (quindi la punizione del colpevole), ma anche rieducativa. Non lo dico io, lo dice la Costituzione.

Non credo che sia frutto della ragione una scelta del genere. Per me, in questo caso, la ragione non è stata per niente interpellata. altro stravolgimento del senso che fornisce il nostro ordinamento giudiziario. Si fa il commissariamento dei centri per migranti. Bene, perché dobbiamo tutelare i crediti dello Stato. Giusto, fate benissimo, d'accordo. Volete tutelarli non dai crediti fiscali - attenzione - ma dai crediti per inadempimenti contrattuali, che non hanno quindi nessun diritto di prelazione. E cosa fate? Accantonate gli utili dell'impresa, perché così lo Stato può fare l'asso pigliatutto, ma vi state dimenticando che esistono altri crediti privilegiati: quelli dei lavoratori che non sono stati pagati. Sono tutelati dal codice civile, non potete stravolgere il nostro ordinamento e le priorità che sono date a crediti più importanti di quelli dello Stato, di gente che lavora e non è stata pagata.

di frustrazione e nell'emarginazione, è chiaro che prima o poi la violenza esploderà. Non state dando sicurezza all'Italia, la state mettendo in una situazione ancora più pericolosa di quella che abbiamo. Rendetevene conto.

orrore nel pensare che uno Stato possa voltare le spalle ai più deboli, quando c'è bisogno di riconoscere i loro diritti umani. provvedimento in esame interviene per mettere ordine sui flussi d'ingresso illegale dei lavoratori stranieri e di prevenzione al contrasto all'immigrazione irregolare, per rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, snellire le procedure per potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti crudeli e criminali degli scafisti. In sostanza, cerca di mettere ordine in tutto ciò che riguarda l'immigrazione clandestina, cosa che la sinistra e i colleghi che mi hanno preceduto non hanno saputo fare quando erano al Governo. un decreto composto da dieci articoli, che intervengono su misure per la programmazione dei flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro. Il decreto interviene altresì su ingresso e soggiorno al di fuori delle quote. disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato e misure straordinarie in materia di gestione dei centri per i migranti e sulla protezione speciale *ex* articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, di fatto una sanatoria illegale. inoltre disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri, argomenti che non vorremmo mai trattare, ma che purtroppo ormai sono all'ordine del giorno e che impegnano continuamente il Governo a trovare soluzioni per evitare morti e stragi. I numeri dei morti sono ritornati a essere esorbitanti e preoccupanti ed è brutto ovviamente attribuire responsabilità su morti e tragedie, ma purtroppo modificare i decreti sicurezza che la Lega aveva fatto ha comportato un aumento incontrollato dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese come dimostrano i numeri. Quando infatti eravamo al Governo ed erano in vigore i decreti di sicurezza di Salvini, nel 2019 gli sbarchi sono stati 11.000, per poi arrivare con le nuove regole a 33.000 nel 2020 e poi a 63.000 e a 105.000 nel 2021 e nel 2022, con un incremento del 60 La strage di Cutro, che ha provocato quasi 100 vittime e che ha avuto naturalmente un grandissimo clamore mediatico, purtroppo non è stata l'ultima. Il primo trimestre del 2023 è stato il più

Il Governo è già intervenuto con il precedente decreto sui flussi migratori a riparare i danni fatti dai provvedimenti adottati dall'ex ministro Lamorgese sullo stravolgimento delle norme d'ingresso che favorivano le ONG, che avevano apertamente e pubblicamente dichiarato di voler violare le leggi italiane. La nostra non è e non è mai stata una posizione di cattiveria, ma l'ennesimo tentativo di cercare di salvare vite umane e tutte queste morti ne sono la dimostrazione. Anche oggi, come tutte le settimane, mi è capitato di sentire il sindaco, il vice sindaco e l'amministrazione di Lampedusa, dove soltanto in questi giorni ci sono stati meno sbarchi, perché c'è stato mare forte, però a Cutro qualche giorno fa è stato un continuo e io, a nome di tutto il Gruppo Lega, voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Lampedusa per essere sempre in trincea e in prima linea con le enormi difficoltà che riscontra. ieri in Commissione ambiente abbiamo avuto l'audizione dell'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Tornando al decreto, un passaggio va fatto sulla protezione speciale, che, come ho già detto prima, rappresenta una sanatoria illegale: non possiamo pensare che si possa fare integrazione semplicemente con il permesso di soggiorno. La protezione speciale rappresenta un fattore attrattivo d'immigrazione di cui il nostro Paese non ha bisogno; è qualcosa che sta mettendo in difficoltà il nostro sistema di sicurezza. È un provvedimento che inoltre garantisce le tutele di chi arriva in Italia e il nostro è un Paese che non deve prendere lezioni da nessuno sulla gestione dell'accoglienza. Noi, però, siamo per un'accoglienza vera, non finta, per un'accoglienza con un'accoglienza con i fatti e non con le parole, quelle di cui la sinistra si è tanto riempita la bocca per poi leggere sui giornali di quattro dei suoi governatori che non hanno firmato lo stato d'emergenza dichiarato dalla Protezione civile e che quindi si sono rifiutati di collaborare nella gestione dell'emergenza. Li vogliono far sbarcare tutti, però poi pretendono che a ospitarli siano altri: questa è la solita ipocrisia rossa. Noi siamo per l'accoglienza, per un'accoglienza giusta che garantisca condizioni di sicurezza idonee e di dignità alle persone che sbarcano. Certamente non saremo mai e poi mai per incrementare quel *business* ghiotto e quelle occasioni di ruberia come quelle che hanno investito recentemente la famiglia Soumahoro. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sottosegretario Molteni, mi si consentirà un fumo di emozione: è la prima volta che parlo in quest'Aula e mi si strozzerebbe la voce in gola se non ricordassi, anche solo per un istante, la memoria del senatore Bruno Astorre mi sembra di sentirlo qui tra noi, con la sua forza terragna, la sua umanità (rara, purtroppo), la sua esperienza che indegnamente proverò a usare come un sestante per cercare orientamento e lume nei mesi che verranno e negli incroci che affronteremo. prendo la parola su un decreto-legge che misura la temperatura di una democrazia come la nostra, ne scruta il senso, ne evoca i fondamenti e ne perimetra i margini, i confini e i bordi. mi rivolgo a loro per il suo tramite, Presidente - oggi non si misura la forza di una maggioranza che si serra, si rinchiude e si blinda - e lo dico senza enfasi - sulla vita delle persone, sulla loro esposta fragilità, sulla loro nudità, sulle loro speranze e sulle loro disperate attese. Proprio questa mattina un ragazzo è morto nel naufragio dello scafo che lo portava a Lampedusa. Era assieme a cinquanta persone - persone, signor Presidente - tra cui undici donne e quattro bambini, che sono state tratte in salvo, come succede ogni giorno che Dio manda in terra. Cambiano i Governi e cambiano le opposizioni, ma non si ferma questo strazio, questo dolore che tutti dovrebbe accomunarci nel rispetto, e invece... Dicevo, signor Presidente, che in quest'Aula oggi non si misura la forza di una maggioranza, ma la qualità di una democrazia, la nostra cultura del diritto, il senso delle cose e l'idea che abbiamo di noi nel mondo. noi nel mondo. Non ho le qualità e le competenze per argomentare con dottrina su questo provvedimento - lo hanno fatto e lo faranno con acribia e puntualità i colleghi - ma desidero sottolineare un punto di fondo più generale e forse vago ma, come si usa dire, politico e che riguarda che razza di Paese Dico "razza" pensando con scorno, per lui e per noi, alle inaccettabili ancorché rivelatrici parole usate ieri da un Ministro, che non nomino per il rispetto che porto per quest'Assemblea e per il Governo del nostro Paese. Incrocio lo sguardo del sottosegretario Molteni, che rispetto molto; perfino mi era parso di scorgere, qualche ora fa, quello del sottosegretario Durigon, che pure dovette lasciare un suo precedente incarico di Governo per l'improvvida proposta di chiamare un parco, intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino, con il nome "Mussolini". Ecco, perfino in lui ho scorto - così mi è sembrato - l'imbarazzo per l'uscita di quel Ministro che non nomino. Dicevo: che razza di Paese emana questo decreto-legge dalla sua lingua di legno, quella che denomina flussi le persone, le donne, gli uomini e i bambini - flussi? - e chiama contrasto l'accoglienza, un'organizzazione intelligente e assennata, civile, torta in uno stato d'emergenza che la dice lunga non sulle questioni di merito, ma sulla paura sì, la paura - che questo Governo e questa maggioranza vogliono evocare, suscitare, alimentare, fomentare e accendere? Colleghi della maggioranza - mi permetterà di rivolgermi a loro, Presidente - la paura che con questo provvedimento volete seminare e piantare nel Paese come un frutto avvelenato, nasce in realtà in voi, vi abita e vi muove fin dai primi passi di questo Governo: la paura dell'altro, del diverso, del non conforme (come si usa dire a destra), dello straniero e dell'estraneo, che, senatrici e senatori, siamo noi, è ognuno di noi. Ciascuno di noi è quell'altro, quel diverso, quel non conforme o quello straniero che credete illusoriamente di fermare, di bloccare e di contrastare. di contrastare, un verbo che, più che dell'altro, dice di voi, rinserrati nella difesa, senza aver compreso cosa abita in voi. Quella paura credete di esorcizzarla proiettandola fuori, additando altrove un nemico, un *bouc un *bouc émissaire*, un capro espiatorio, per non realizzare e confessare quello che la paura che fa e che mette questo decreto-legge dice di voi. La paura degli italiani si legge nel provvedimento in discussione. Una sfiducia profonda nei confronti di questo Paese, della sua capacità di accogliere e integrare e di crescere insieme, come si fa - badate non in un irenico mondo ideale, ma nel resto del mondo; di sicuro, nel resto d'Europa. Governare con la paura, come sa chi va per mare e governa la sua imbarcazione (in senso etimologico), ma punta in verità al naufragio, lo cerca. Dicevano gli antichi: *naufragium feci, bene navigavi*. Questo cortocircuito logico è esattamente la fallacia del vostro provvedimento, al quale noi oggi qui, questo sì, ci opponiamo, con una forza che viene dalla passione per ciò che è fragile, per l'umano e per le persone, che è un altro modo di dire la politica, il suo senso e il suo orizzonte. Per non guardare quei volti - sì, senatrice Minasi - per non sentire le loro storie, per non ascoltare la loro sete di futuro, li sterilizzate in questa neolingua che marcisce in gola e che spersonalizza, secondo una movenza che è non solo della nostra burocrazia, ma anche della destra, che, per la complessità della sua storia, utilizza sempre questo doppio registro: non dico, ma evoco (e noi altri ci siamo intesi). Trovo in questa ipocrisia, quella dei flussi e del contrasto, la pellagra di chi non ha il coraggio di dire ciò che suggerisce, la strizzata d'occhio, il segnale convenuto, il "capisci a me". Se avete il coraggio, ditelo; ditelo qui, in quest'Aula, cos'avete in mente con questo provvedimento. Ditelo senza infingimenti, circonlocuzioni, esoterismi. Santo cielo, la sostituzione etnica, le palette identitarie! Ditelo, come avete fatto in piazza nei vostri raduni. C'è abbondanza di immagini sulla Rete, con la sicumera dell'opposizione degli anni scorsi, già oggi anche della mia. della mia. La rassegna stampa sarebbe efficacissima, ma io non cerco una *clip* da condividere sui *social*, quanto piuttosto un filo di ragionamento comune. Argomenti quadrati e testardi sono stati richiamati a più riprese oggi in Aula: i numeri veri dei migranti, l'allarme dei sindaci e delle comunità, le preoccupazioni di chi fa impresa. Eppure, sottosegretario Molteni, dovrebbero premervi i timori delle ONG e delle associazioni, il grido della Chiesa, i profili di costituzionalità, il quadro normativo europeo, e potrei continuare. Argomenti che fanno ballare i gangheri del vostro decreto-legge e lo smontano agli occhi dei cittadini, che - badate bene cercano verità e chiarezza, motivazioni ben fondate e non capestri, perché è su questa solidità che si costruiscono le comunità e il nostro stare assieme, non sui vostri spettri, su parole d'ordine fuori tempo e fuori sincrono, sulla faccia feroce. Guardate non risponde ai problemi questa vostra tetra *haka*. Signor Presidente, in conclusione, chiedo: ma con la corsa che il Paese tutto è chiamato a fare sul PNRR, su un'occasione irripetibile di sviluppo e di riforma del Paese, che il Governo sta trattando come se i soldi li dovessimo cacciare noi e non ce li dessero, vi pare che stiamo qui a discutere se la protezione speciale porti più o meno persone in Italia o se il problema della denatalità si affronta agitando il piano Kalergi? A noi così non pare ed è per questo che non concludo questo intervento con l'invito al Governo e alla maggioranza a fermarsi, perché a fermarvi non saranno la vostra coscienza o la nostra opposizione in quest'Aula, temo, ma i fatti. Sarà la durezza sconveniente della realtà a sconfessare questa ideologia, questa crudeltà sottovuoto; sarà la vostra paura, quella che pensavate di far germogliare tra la gente, che in realtà vi assilla e vi tormenta, a far tremare quello che avete portato in Aula.

Lollobrigida: forse noi avremo paura del diverso, ma mi sembra che voi abbiate un po' paura del vocabolario italiano. *(Applausi)*. Ad ogni buon conto, credo che questo Governo, in cinque mesi, abbia dispiegato tutto quello che poteva dispiegare in poco tempo e che stia facendo di tutto per fermare l'immigrazione clandestina e gli sbarchi, quindi per favorire la diminuzione delle morti nel mar Mediterraneo: tre decreti, tutti e tre citati meglio di me dai colleghi, accordi bilaterali con i Paesi frontalieri per attuare il piano Mattei e con l'Africa, visione in Europa

stilato un accordo con Sunak per difendere i confini della Manica dall'immigrazione e che saranno schierati centinaia di agenti per difendere i confini dall'immigrazione clandestina. D'altro canto, e manterremo un impegno costante, nella consapevolezza che esiste un problema e nella consapevolezza del nostro obiettivo, che è quello di bloccare le partenze, rimpatriare gli immigrati immigrati clandestini che sono venuti in Italia e integrare gli immigrati che ne hanno diritto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo. Non abbiamo capito francamente quale sia il vostro. E lo dico perché è è curioso vedere come la sinistra, in generale, abbia sempre la capacità di schierarsi esattamente dalla parte opposta rispetto agli interessi dell'Italia e degli italiani. non è che risolve i problemi. Quando ci sono problemi, la sinistra trova sempre il modo di girarsi dall'altra parte per non guardarli e di alzare bandiera bianca di fronte ad essi (a volte forse più la bandiera rossa). Sono queste le soluzioni che state proponendo all'Italia. C'è il problema degli anarchici, di Cospito, del 41-*bis*? Togliamogli il 41-*bis*, che problema c'è? C'è il problema della droga e dello spaccio? Legalizziamo le droghe, che problema c'è? C'è il problema dell'immigrazione clandestina? Saniamo tutti i clandestini, prendiamoli tutti, facciamoli venire in Italia e diamo a tutti un permesso di soggiorno, saniamo quelli che sono già clandestini; gli diamo la cittadinanza con lo *ius soli* e abbiamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina (non ci sono più clandestini, d'altro canto). Noi abbiamo un'altra visione, ci dispiace, fatevene una ragione. Noi non ci volteremo dall'altra parte: vogliamo fare di tutto per bloccare gli sbarchi e per risolvere il problema, che non riguarda soltanto quelle persone, ma gli italiani. Gli sbarchi vanno fermati: è molto semplice, è banale. Capisco che, tutte le volte che si parla d'immigrazione, voi utilizzate la retorica che gli immigrati ci servono; gli immigrati ci servono per risolvere tutti i problemi che abbiamo in Italia. Non facciamo più figli? Ci servono gli immigrati, li fanno loro. Servono lavoratori? Non c'è problema, servono gli immigrati per il lavoro italiano. qualsiasi problema, per qualsiasi cosa che non fanno più gli italiani, la soluzione è: la fanno gli immigrati. Anche votare PD: non lo fanno più gli italiani, probabilmente domani lo faranno gli immigrati. *(Applausi. La nostra è una soluzione molto diversa. Molto banalmente, se c'è un problema di denatalità, vogliamo risolvere il problema della denatalità; vogliamo aiutare le mamme a fare figli promuovendo politiche di conciliazione con il lavoro, vogliamo premiare le famiglie, cosa che faremo con l'azione di Governo.

non pensiamo che si risolva solo con gli immigrati. È una delle ragioni per le quali vogliamo togliere il reddito di cittadinanza, per far andare a lavorare anche i cittadini italiani che possono farlo, che sono occupabili e che domani dovranno andare a lavorare. O vogliamo risolvere tutto con gli immigrati? Sono curiose questa retorica e questa narrativa della sinistra, secondo cui voi state con i poveri e con le persone che hanno bisogno, mentre noi siamo brutti, cattivi e disumani. Però poi è bello vedere come la mattina vi fate un giro per le Caritas, magari nelle ONG, e la sera i vostri *leader* di partito fanno le cene di gala negli attici di cantanti famosi, con Jovanotti e altri, mangiando caviale e godendosela. *(Applausi)*. È un po' curiosa questa cosa, no?

è far arrivare quelle persone e lasciarle in mezzo a una strada. Disumano è lasciarle nelle mani della criminalità, perché più persone vengono, più morti in mare ci sono o più criminalità c'è nel nostro Paese, perché queste persone finiscono costantemente nelle mani della criminalità: basta accendere un telegiornale per vederlo. vederlo. Disumane sono quindi le proposte che fate: quelle, sì, sono disumane. L'immigrazione clandestina è un problema e ne siamo consapevoli; è un problema che va risolto, per l'Italia, per gli italiani e anche per quelle stesse persone. Quindi, mettetevi il cuore in pace. mettetevi il cuore in pace. Forse i dati e i numeri oggi non ci danno ragione, ma gli italiani sanno che questo problema lo vogliamo risolvere. Gli italiani sanno che i confini li difendiamo sempre, non quando ci pare. Non è che i confini ci sono solo tra l'Ungheria o tra la Russia e l'Ucraina: e l'Ucraina: ci sono anche in Italia e in Europa e vanno difesi dappertutto. È per questo che non ci arrenderemo, fatevene una ragione. È per questo che credo che gli italiani siano più sereni che ci sia il centrodestra a governare e che ci sia Giorgia Meloni al Governo perché, se non ci fosse Giorgia Meloni, oggi forse gli sbarchi sarebbero il doppio, il triplo o il quadruplo.

cui dire di no dimostra un'insensibilità del Governo verso i valori condivisi dalla nostra Nazione. Poteva essere invece l'occasione per dimostrare che c'è umanità, che c'è sensibilità, che c'è empatia, anche quando si ha a che fare con il freddo costrutto normativo.

Presidente, sono universali e non riservati soltanto alla comunità italiana. La legge italiana vale per tutti, si applica sul territorio italiano. Oppure i vostri valori della famiglia sono quelli, non soltanto della famiglia tradizionale, ma della famiglia italiana? Vi rivolgo questa domanda.

linguale. Voi state promettendo agli italiani un clima di sicurezza. Ma, se non favoriamo le politiche di integrazione, voi state andando nella direzione opposta. Rischiamo di creare emarginazione, rischiamo di creare tensioni sociali.

Scalfarotto, esaminando dicono più o meno la stessa cosa. Essi dicono sostanzialmente che i lavoratori stranieri che sono in Italia e hanno un contratto di lavoro devono essere regolari, devono essere regolarizzati. Non ha senso avere persone che hanno dei lavori (perché i nostri imprenditori hanno bisogno di loro) e noi legislatori le lasciamo in uno stato di irregolarità. *(Applausi)*. Ciò vuol dire che queste persone avranno meno diritti; vuol dire che queste persone naturalmente saranno più a rischio dal punto di vista sociale e della marginalità; vuol dire di conseguenza che queste norme servono a garantire quella sicurezza di cui questa maggioranza si fa portavoce. Allora, se noi abbiamo delle persone, come è successo recentemente durante il *click day*, con 80.000 posti messi a disposizione 240.000 richieste, la domanda è, cari colleghi: i 160.000 che avevano pronti i contratti di lavoro e i cui datori di lavoro hanno chiesto la regolarizzazione, perché ne avevano bisogno, mi dite che cosa saranno, se non 160.000 irregolari che abbiamo nel Paese e che voi avete reso irregolari? *(Applausi)*. Sarebbero persone che hanno un lavoro in questo nostro Paese. E allora chiedo come si fa a non votare emendamenti di questo genere. Qui c'è una responsabilità molto precisa da parte vostra, perché - ripeto - sono persone di cui le nostre famiglie hanno bisogno. Magari si tratta di badanti, di persone che hanno la cura dei componenti si tratta di lavoratori agricoli, si tratta di lavoratori del turismo, si tratta di tutte quelle persone che le nostre associazioni datoriali, a partire da Confindustria fino a tutte le altre, ci chiedono di regolarizzare. I pareri del Governo del Governo sono irrazionali, che danno l'impressione - è soltanto un'impressione, sottosegretario Molteni - che vogliate promuovere l'irregolarità. Quell'irregolarità impedisce che la vicenda strategica, epocale, strutturale delle migrazioni venga gestita in modo razionale, con un approccio di lungo periodo,

vicenda razionale - non avremmo più l'allarme sociale che avete pompato negli ultimi anni. Chiedo quindi, ovviamente, agli altri Gruppi di opposizione di votare l'emendamento a mia prima firma, come tutti quelli che stiamo votando, ma devo sottolineare davanti alla pubblica opinione e al Paese, che stanno seguendo i lavori,

il numero delle persone irregolari e garantire, specialmente a coloro che già lavorano o già hanno dato prova di una effettiva integrazione nel Paese, di acquisire un titolo di regolarità permanente. Mi lasci dire, signor Presidente, che è davvero inspiegabile il fatto che il Governo si ostini a dare parere negativo. Abbiamo presentato una serie di emendamenti per rendere possibile un processo di emersione dal lavoro nero e per rendere quindi possibile l'inserimento regolare nel sistema produttivo del nostro Paese. L'unica risposta che abbiamo ricevuto a questi emendamenti è stata l'insistenza nel formulare in maniera ancora peggiorativa l'articolo 7, di cui diremo in seguito, che ha anch'esso - esattamente come il parere negativo a questi emendamenti - l'unico effetto di aumentare il numero della presenza irregolare nel nostro Paese, con danno per tutti. Ciò è infatti un danno, naturalmente, per gli interessati, che non potranno partecipare in maniera regolare al nostro sistema produttivo, e un danno per tutte le nostre imprese e tutti i nostri concittadini.

anche su quelli immediatamente successivi, come l'emendamento 2.12, a mia prima firma, o quelli di cui parlava adesso l'onorevole Giorgis, perché sono tutti più o meno relativi alla stessa materia e tutti insistono sullo stesso tema. sullo stesso tema. In questi giorni, in Commissione, siamo stati molte ore e molti giorni a discutere e a proporre emendamenti che davvero ci sembravano di puro buonsenso e che

non a ridurre l'irregolarità, ma ad aumentarla? La ragione me la sono chiesta, in questi giorni. Anche io non ho capito il motivo per cui arrivava sempre un parere negativo. Certamente mi ero dato una risposta, ma poi nella giornata di ieri ho compreso che quella mia risposta era parziale. La risposta che mi ero dato era molto semplice, cioè che in qualche modo

un argomento di campagna elettorale, quello che viene usato sempre per prendere i voti, per avere consenso e perché in qualche modo, attraverso quel tipo di argomento

leggo invece da parte di autorevolissimi esponenti della maggioranza la tesi classica del suprematismo, cioè la tesi della sostituzione etnica, allora capisco. Capisco il motivo per cui a tutti questi emendamenti di buonsenso è stato ripetutamente detto di no. Concludo, Presidente,

cioè la sostituzione di chi evidentemente non sa fare il suo lavoro, pensa di governare il Paese continuando a fare propaganda, è abituato a prendere i voti semplicemente alimentando le peggiori paure e i peggiori istinti di questo Paese e secondo me non è degno e non merita di governare l'Italia.

Presidente, lei giustamente ha eccepito l'irritualità di un Gruppo che esprime un parere e poi lo rinnega in Aula, come ha fatto prima. Io però esprimo un po' di perplessità sul fatto che il Governo continua a pareri su emendamenti ufficialmente ritirati (e ce ne sono sei o sette a ogni articolo). Chiedo quindi che il Governo aggiorni il suo fascicolo, perché esprimere pareri su emendamenti ufficialmente ritirati per l'Aula crea un po' di confusione rispetto alle votazioni.

connesso alla questione dei flussi migratori, ma è un aspetto un po' tecnico legato al settore marittimo. Sostanzialmente, le imprese del settore marittimo ci hanno segnalato ha avuto anche una certa visibilità sugli organi di stampa - che con la normativa che abbiamo attualmente, i lavoratori extracomunitari che lavorino su una nave che attracca in un porto italiano, per esempio sulle navi da crociera (sapete che molti lavoratori delle nostre imprese, anche crocieristiche, vengono da altri Paesi), nel momento in cui la nave arriva in porto dovrebbero essere scaricati, messi su un aereo e rimandati immediatamente nel Paese di provenienza, il che provocherebbe notevoli problemi operativi a quelle vere vere e proprie città galleggianti che sono le nostre navi da crociera, ma anche su più piccole imbarcazioni. Allora, noi abbiamo cercato, con questo emendamento, di allargare l'ipotesi del permesso di soggiorno e del visto che si ha quando la nave è ormeggiata nel nostro Paese ad altre situazioni, quindi anche quando la nave sia in transito, sia in arrivo o in partenza.

non ha a che fare immediatamente con i flussi migratori generalmente intesi, ma con una fattispecie molto specifica che però riguarda moltissimo la nostra nautica, che - come sapete - è uno dei settori di massima eccellenza del nostro *export* e del nostro *made in Italy*. Chiederei, se possibile, al Governo di accantonare questo emendamento per verificare, magari con gli uffici, se tecnicamente questa cosa abbia senso, perché - ripeto - non va a incidere immediatamente sul grande fenomeno dei flussi migratori, ma va ad incidere su un settore del *made in Italy* importante, come la nostra nautica, e del turismo, come la nautica da diporto e la nautica crocieristica, per cui potremmo utilizzare questo particolare veicolo legislativo per risolvere un problema che sembra riguardare magari una minoranza, un piccolo gruppo, però è un gruppo molto importante per la nostra economia. Chiederei al Governo di cambiare parere. Mi rendo conto che farlo in corsa non è però se il sottosegretario Molteni volesse acconsentire all'accantonamento e approfondire la questione con gli uffici, gliene sarei grato soprattutto a nome delle imprese della nautica e della crocieristica, che sono appunto molto importanti per il nostro Paese.

parere contrario

e del voto che esprimeremo. L'emendamento 5.0.100/6 cerca di ovviare al tentativo di ancorare la sostanza dell'emergenza, ossia le deroghe alla normativa vigente con i poteri speciali

Formalmente l'emergenza dichiarata potrebbe anche decadere, ma di fatto le deroghe che essa istituisce permangono attraverso il decreto-legge. Il nostro emendamento fa in modo che invece le deroghe siano ancorate alla durata dell'emergenza.

capisco che la normazione dell'emergenza possa giustificare delle deroghe. Sono un giurista e so bene che, in alcuni ambiti, ci sono delle differenze e che questo può consentire tutto. Finché si tratta di snellire procedimenti burocratici e di favorire una velocizzazione, sono ammesse tutte le deroghe del mondo, ma non senza limiti. Questo emendamento vuole sottolineare l'importanza, comunque, di garantire almeno la tutela ambientale, la tutela paesaggistica, soprattutto delle nostre coste, e la tutela dei beni culturali. Quindi, non capisco il parere contrario del Governo. Forse non avete a cuore questa ricchezza, che è del popolo italiano. Ricordate, infatti, che la qualità della vita si basa anche sulla possibilità di godere di quello che è un bene comune di tutti noi. Le linee politiche del Governo spesso non sembrano così sensibili alla tutela ambientale, invece il MoVimento 5 Stelle vuole la tutela ambientale, non soltanto per rispettare i diritti e le aspettative degli italiani di oggi, ma anche quelli delle prossime generazioni.

questo emendamento dice che le donne vittime di violenza, per le quali è stato accertato che siano state vittime di violenza, vengono trasferite, in via prioritaria, presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale. Ora io vorrei capire - già ci ho provato in Commissione, ma non ho avuto una risposta - per quale motivo la maggioranza si oppone a una misura così sensata, a tutelare le donne vittime di violenza inviandole presso i centri dove possono essere accolte e sostenute. Senatore Scalfarotto, il suo Gruppo avrebbe terminato il tempo a disposizione. Eccezionalmente le do due minuti, però mi sembrano utilizzati particolarmente bene in questo caso, visto che ci stiamo occupando di vittime di violenza e che quest'Aula in più occasioni ha avuto l'opportunità di esprimere la propria condanna di questo tipo di violenze di violenze perpetrate nei confronti delle donne. Si tratta di evitare un automatismo. Non dobbiamo trattare queste persone come se fossero pacchi postali; in particolare, quando ci sono particolari circostanze di debolezza o di fragilità, credo che il legislatore dovrebbe avere la civiltà e la coscienza di occuparsi di queste persone, come per esempio le donne vittime di violenza. Negli emendamenti già respinti abbiamo parlato di persone vittime di tortura, di persone LGBT e di tutta una serie di categorie di persone che sono particolarmente gravate, oltre che dal viaggio, dalle torture, dalle difficoltà e dalla traversata, anche da problemi ulteriori, sui quali quest'Aula molto spesso ha espresso la sua condanna. Quindi direi che è coerente da parte nostra votare a favore di questo emendamento

Mi appello di nuovo alla sensibilità umana di questo Governo, perché vede, Presidente, i migranti non sono cose, non possiamo considerarli carichi residuali: sono persone. E se credete nel valore della famiglia, dimostratelo anche quando vi occupate della normazione.

le farò perdere solo pochi minuti, perché ha dell'incredibile questo parere negativo. Probabilmente non avete letto il testo, così come penso che non abbiate letto il testo del precedente emendamento, che è stato respinto. Non tenere conto, nella determinazione dei criteri di riallocazione delle persone trattenute nei centri di prima accoglienza, dell'unità dei nuclei familiari, o non tenere conto dei minori che devono rimanere ovviamente insieme ai genitori, lasciatemi dire

necessario respingere un emendamento che si limita a esplicitare il principio in base al quale i nuclei familiari non vanno smembrati e i minori devono comunque rimanere insieme ai genitori. Quale sarebbe il danno dall'accogliere questi emendamenti? Mi chiedo, se questi emendamenti venissero accolti, quale sarebbe, secondo il Governo e la maggioranza, il danno che questo vostro legiferare produrrebbe. Chiedo scusa all'onorevole collega che si lamentava del fatto che non ho alzato la mano immediatamente, ma l'Assemblea può permettersi di far passare senza spendere una sola parola un voto che nega questo elementare principio?

perché vorrei, attraverso la Presidenza, comunicare al collega Giorgis che è già così.

di essere accolte da qualche operatore che sappia capire la loro condizione. Si tratta molto spesso di donne che non solo non sono consapevoli dei propri diritti, ma che fanno fatica a raccontare o addirittura a raccontare o addirittura ad essere consapevoli di quello che hanno subito e che tante volte sono addirittura accompagnate dagli uomini che hanno esercitato su di loro violenza, tanto nel Paese d'origine, quanto nei lunghi viaggi che sono state costrette a percorrere. Quindi, è proprio indispensabile come abbiamo detto al sottosegretario Molteni, anche in applicazione del principio che nel suo emendamento il Governo ha provato ad affermare. In Commissione glielo abbiamo ripetuto più di una volta: l'emendamento del Governo è stato giustificato dal sottosegretario Molteni, a più riprese, che era sostanzialmente volto a rendere più compatibile il sistema con il rispetto della dignità delle persone, perché favoriva dei numeri più sostenibili nei centri di prima accoglienza.

qualche modo, anche una volontà espressa, ma secondo noi non inverata, nell'attività del Governo e negli atti che ha messo in campo. Noi vi diciamo: mettete nei centri di prima accoglienza operatori e operatrici in grado di capire se quella donna effettivamente ha subito violenza,

a favorire percorsi di integrazione e, se l'integrazione per noi è la parola maestra da perseguire, questa è una condizione essenziale anche eventualmente per favorire poi il passaggio delle donne delle donne nei centri antiviolenza (CAV), di cui all'articolo che abbiamo chiesto prima di accantonare. Chiederei, quindi, se abbiamo accantonato quello precedente, di accantonare anche questo e di provare in qualche modo almeno a riscrivere un emendamento che abbia un senso e che provi veramente a salvaguardare i percorsi di donne che hanno già subito delle sofferenze tanto atroci e alle quali forse andrebbe evitato un ulteriore percorso di sofferenza. Signor Presidente, come abbiamo già spiegato in Commissione e ha detto molto succintamente il senatore Balboni, tutti questi emendamenti propongono una serie di attività che vengono già svolte,

anche da tante associazioni di volontariato che svolgono proprio i servizi che vengono qui proposti, compreso quello di tutelare le donne e i minori, di non separare le donne dai minori. Sono tutti i servizi che oggi come ieri vengono erogati all'interno dei centri di accoglienza. Votare questi emendamenti non vuol dire altro che affermare che fino ad oggi queste attività, le nostre associazioni di volontariato, lo Stato, le associazioni che sono coinvolte non le hanno svolte e ammettere che questo non avverrebbe. Se voi avete contezza che ciò non avviene, non avviene, denunciatelo pubblicamente; diversamente votare questi emendamenti vorrebbe dire mettere una croce sulle tante attività di volontariato che ha svolto lo Stato e che hanno svolto le associazioni ed è una delle ragioni per le quali

ho chiesto la parola perché penso che sia necessario sostenere queste emendamento e sostenerlo con una logica che deve essere molto chiara: noi non possiamo lasciare queste attività ad una iniziativa volontaristica. Noi abbiamo il dovere di organizzare questo servizio perché sappiamo perfettamente che possono esserci casi, anche numerosi, di donne oggetto di violenza *(Applausi)*. E il fatto di imporre in una legge una previsione circostanziata obbliga

personale, quello che c'è già e gli eventuali costi che devono essere messi in campo. Altrimenti diventa un emendamento un po' strumentale per dire abbiamo detto di no, così andate a dire ai cittadini che abbiamo detto di no a un intervento per cercare di mettere in campo azioni per tutelare le donne che sono state vittime di violenza. Io penso che sarebbe più corretto fare questo tipo di intervento. È un tema che si può porre, che si porrà in un'altra occasione, ma occorre un approfondimento, uno studio relativo a quello che succede oggi. È infatti possibile che magari già lo Stato paghi un servizio - come sicuramente sarà per le donne vittime di violenza e sarebbe quasi come squalificare quel servizio a favore qualcosa che non sappiamo se sarà disponibile o meno. Le cose si fanno con intelligenza, soprattutto quando si tratta di argomenti seri. Pertanto, dico che sensibilità sul tema c'è, lo approfondiamo e magari lavoreremo a un disegno di legge o a un emendamento su un prossimo decreto-legge, perché poi bisogna quantificare anche il costo, bisogna tornare in 5a Commissione, valutare anche la disponibilità dei centri antiviolenza e vedere quanti ce ne sono. Ad esempio, ricordo che già si denunciava una mancanza di personale per affrontare tutte le denunce che vengono fatte. Si tratterebbe, quindi, di un potenziamento dei centri antiviolenza a livello generale; sono tutti elementi che vanno valutati, non possiamo farlo in Aula con un emendamento che altrimenti rischia solo di essere strumentale. Io prima ho sentito tutte le vostre proposte: facciamo emergere tutto il lavoro nero che c'è.

l'emendamento 5.0.100/50 interviene su una disposizione normativa che attribuisce al prefetto la possibilità di ospitare i migranti in strutture provvisorie. Tuttavia, non dà una definizione temporale. C'è un inciso - ed è qui che vogliamo intervenire - che dice «per il tempo strettamente necessario». Signor Presidente, quanto è il tempo strettamente necessario? Un anno, sei mesi, sette giorni? Vogliamo dare un po' più di certezza di diritto? Queste formulazioni non sono in linea con la tecnica normativa,

faccio presente che c'è un parere contrario da parte della 5a Commissione. Presumo che ci sia quindi una valutazione di impatto economico, qualora l'emendamento venisse preso in considerazione. alla luce dell'importanza di una valutazione ulteriore, che potrà essere fatta successivamente, senza però tralasciare l'importanza del tema che è stato sollevato dalle opposizioni, che ha trovato un un riscontro positivo anche da parte della maggioranza e una valutazione di grande attenzione da parte del Governo, inviterei i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in modo tale che rimanga un impegno nei confronti del Governo a riproporre il tema in uno dei prossimi provvedimenti, facendo anche una valutazione ulteriore e più ampia per capire se questo servizio oggi viene o non viene garantito all'interno dei centri, a tutela delle donne vittime di violenza ed eventualmente di prendere in considerazione l'ipotesi di inserirlo in un futuro provvedimento.

a vantaggio delle donne vittime di violenza. Naturalmente avremmo preferito che il parere fosse favorevole sull'emendamento e che questa misura potesse essere inserita in

che, per certi versi, gli immigrati sono anche una risorsa. Lo avete capito, perché ve lo chiede il mondo dell'imprenditoria. Adesso ditemi perché: onorevoli colleghi, come avete stabilito che le quote, per il 2023, debbano essere di 80.000 unità.

sono insufficienti a dare risposta alle esigenze produttive. Allora vi chiedo se tenete o meno al sistema produttivo italiano, perché in questo modo rischiate di danneggiare gli imprenditori italiani.

che supponiamo siano sensibili al tema di una buona relazione con i sindaci e i Presidenti delle Regioni, sul fatto che questo articolo manomette davvero il sistema dell'accoglienza e priva i sindaci e i Presidenti delle Regioni della possibilità di pianificare, di gestire e di affrontare il tema,

più di così, che è ingestibile e che non si può calare sulle loro teste un problema che diventerà ancora più grande? Cosa dobbiamo immaginare? Voi ci assicurate che non ci saranno le tende, come se tutto il problema girasse intorno alle tende. Il tema se staranno nelle tende - il che, semmai, apre un problema di difesa dei diritti umani - o se staranno nelle caserme dismesse o se verranno individuati luoghi che i sindaci dovranno vedersi evidentemente imposti, che sarà il prefetto a scegliere. Questo davvero colpisce, in particolare se si pensa alla dottrina sulla quale la Lega in questi anni ha Lega in questi anni ha costruito il proprio consenso politico, che è di una buona relazione con il territorio e con gli enti locali. Non è così che si può produrre qualcosa di buono.

un problema che voi dite di sicurezza e che noi invece sosteniamo essere più razionale, cioè di buona gestione, di integrazione, che necessiterebbe di fare un passo avanti nella buona relazione tra i cittadini e gli stranieri che arrivano. Voi mettete davvero i sindaci in enorme difficoltà e io credo che questo si rivelerà subito. Non ci sarà bisogno Non ci sarà bisogno di aspettare molto per vedere i cattivi risultati di questa decisione. Abbiamo tentato, in Commissione, di ragionare su questo

al secondo periodo, le parole: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale».

L'emendamento 6.5 interviene su una disposizione normativa che prevede il commissariamento dei centri per i migranti quando sono inadempienti nei confronti dello Stato;

dall'articolo 2751-*bis* del codice civile. Ci sono lavoratori che non hanno percepito lo stipendio e lo Stato prende tutto e lascia in bianco i lavoratori.

Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione. Vorrei anche dire due parole su questo ordine del giorno, a cui tengo molto. L'avevo spiegato in Commissione: questo ordine del giorno è semplicissimo e chiede di fare chiarezza, in particolare in favore degli enti locali, sui contributi statali ed europei che ci sono per garantire l'integrazione dei cittadini regolarmente residenti nel nostro territorio, con un occhio di riguardo per le donne e i giovani, i minori in generale e i bambini, perché da sindaco ho notato che ultimamente, probabilmente anche perché siamo sempre alle prese con qualche emergenza, purtroppo stanno arrivando meno informazioni ai territori, anche da parte di associazioni e cooperative, riguardo a come utilizzare i fondi che ci sono. Quindi, non si chiedono soldi in più, perché i soldi ci sono e sono anche tanti (ricordo per esempio il integrazione, che è forse il più noto di tutti), però spesso non arrivano le informazioni nei Comuni: parlo di soldi che servono per fare i corsi di lingua, in particolare per le donne ma non solo, o per l'integrazione dei giovani e spesso si devono utilizzare risorse che per fortuna nei nostri territori

garantire una migliore integrazione. Ne parliamo sempre tutti, però parlarne non basta più. Bisogna integrare i cittadini regolarmente residenti nel nostro Paese.

vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e anche del Governo su questo emendamento, che sta per essere messo in votazione, e vorrei che vi fosse piena consapevolezza di cosa quest'Aula sta per votare. L'emendamento è molto semplice: esso prevede la abrogazione di una parte dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina le modalità di trattenimento e di accoglienza. L'articolo 10,

anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e la somministrazione di corsi di lingua italiana e servizio di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui agli articoli successivi. abbiamo una legge dello Stato che prevede espressamente che siano assicurati, a coloro che sono trattenuti nei centri di prima accoglienza, oltre ai più elementari ed essenziali beni materiali, anche la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. L'emendamento che stiamo per approvare chiede di sopprimere di sopprimere questa parte dell'articolo 10 della legge n. 142 del 2015 e quindi di far venir meno, tra le prestazioni e i servizi assicurati a coloro che sono trattenuti, la la mediazione linguistico-culturale. Noi riteniamo che non sia più necessario garantire, a coloro che tratteniamo, quel minimo livello di capacità di comprendere la loro situazione e non siamo più neanche disponibili a consentire loro di avere contezza dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso i servizi di orientamento legale. servizi e condizioni essenziali che dal 2015 faticosamente tentiamo di garantire. Presidente, Presidente, per il suo tramite chiedo al Governo o a qualche esponente della maggioranza di alzarsi in piedi, di prendere la parola e di dire a quest'Aula perché bisognerebbe eliminare questi essenziali servizi.

all'interrogativo del senatore Giorgis, che secondo me è molto pertinente, mi permetto di rispondere io al senatore Giorgis, perché credo di sapere le ragioni per cui, anche se sembra incredibile, viene presentato un emendamento come questo. E sa la ragione qual è, Presidente? Queste cose, senatore Giorgis, costano qualche soldo, qualche piccola risorsa. Evidentemente si pensa di poter fare a meno di essenziali situazioni e di mettere per l'appunto i migranti in una condizione ancora più difficile di quella in cui sono. Ricordiamoci sempre che parliamo di prima accoglienza, di persone che arrivano di persone che arrivano da viaggi drammatici e da condizioni drammatiche. Evidentemente si risparmia qualche centesimo sulla pelle di quelle persone, esattamente mentre - come sappiamo si aumentano le spese militari e si fanno cose che vanno in una direzione completamente diversa. È questa la ragione, senatore Giorgis.

all'emendamento 7.301, che interviene su aspetti importanti, come la cancellazione delle condizioni psicofisiche o di altre motivazioni, che spesso sono servite

a parte l'irritualità della procedura, è interessante del presentatore di un emendamento che per settimane è stato su tutte le cronache - è questo l'emendamento di cui si è parlato per settimane - e sul quale il Governo, in Commissione,

che proponeva originariamente, dell'inciso: «,o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6». Quali sono, onorevoli colleghi, gli obblighi di cui all'articolo 5,

*(Applausi)*. Dunque vorremmo che, in questa irritualità, il senatore Gasparri ci spiegasse, insieme a tutta la maggioranza, perché l'emendamento è sottoscritto non solo dal senatore Gasparri, ma da senatori di tutta la maggioranza, se questo ravvedimento dell'ultimo momento è operoso, che alla fine, come sarebbe saggio, indurrà il sottosegretario Molteni ad alzarsi, fra poco, e a dire che anche l'emendamento del Governo, che forse in maniera abbastanza controversa, vuole abrogare la protezione speciale, in realtà verrà ritirato. Delle due l'una: o lo avete presentato temendo che il richiamo al rispetto degli obblighi internazionali, alla Carta di Nizza e alla CEDU imponga al nostro Paese di continuare a garantire la protezione speciale avete capito che a questi obblighi non possiamo sottrarci e non possiamo farlo non solo perché - come è stato specificato nella nota del Quirinale che ha accompagnato l'approvazione del decreto - noi agli obblighi internazionali non vogliamo e non dobbiamo sottrarci *(Applausi)*, ma anche perché forse vi siete resi conto - voglio sperare - che eliminare la protezione speciale avrà come unica, quella di aprire un contenzioso infinito. Gli obblighi internazionali permangono e, quindi, potranno fare ricorso e chiedere l'applicazione della Carta di Nizza e della CEDU. Forse, sarebbe bene quindi ridurre l'incertezza, ridurre il rischio di irregolarità e rinunciare a questo decreto o perlomeno all'articolo 7.

Signor Presidente, siamo arrivati al cuore del provvedimento e non possiamo che sottolineare che le questioni pregiudiziali di costituzionalità che avevamo fatto valere questa mattina adesso vengono al pettine. Questo è il tema. È un ravvedimento operoso? È un'indicazione che ci viene dalla saggezza di chi aveva già detto, quando avete chiesto l'abolizione della protezione umanitaria, della protezione umanitaria, che gli obblighi internazionali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali non potevano essere violati? Ci siamo arrivati?

speciale. Questo è il punto. *(Applausi)*. Fermatevi voi, prima che ve lo dicano i giudici della Corte costituzionale e i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea.

illustrato dai senatori Giorgis e Lombardo. Credo che sia del tutto illegittimo che un senatore riformuli un proprio emendamento,

Altrimenti, su ogni emendamento possiamo proporre riformulazioni e avere il parere del Governo. Credo che sarebbe stato più logico chiedere prima l'espressione del Governo, che casomai avrebbe potuto riformularlo nella direzione che che il presidente Gasparri ha voluto indicare all'Assemblea. Ma questo diventa un precedente che io ritengo sia difficile da gestire nelle settimane che verranno.

come se la protezione speciale non esistesse più dall'oggi al domani con l'arrivo di questo provvedimento e col nostro emendamento. In realtà, la protezione speciale si chiama in quel modo per casi speciali ed eccezionali, probabilmente sarebbe stata chiamata protezione normale, protezione a tutti, salvaguardia per tutti e quant'altro. Noi abbiamo cancellato l'estensione

non ho interrotto e non ho fatto rumore sulle vostre dichiarazioni. Dico semplicemente che ci manca solo che facciamo una norma che viola il diritto comunitario o le norme internazionali.

previste dal diritto internazionale sono il diritto d'asilo, se scappano dalla guerra, e la protezione sussidiaria, se il ritorno in patria costituisce per loro grave pericolo; naturalmente il diritto comunitario afferma che ogni Stato può mettere in campo delle forme di protezione complementare. Prima c'era la protezione umanitaria,

signor Presidente, andare a verificare effettivamente le condizioni psicofisiche dell'immigrato che arriva e con questa scusa molti hanno ottenuto sostanzialmente la protezione speciale. in Aula).* Se non avete timore di quello che dico, non interrompetemi. L'altra questione riguardava un'altra dicitura che è stata introdotta, quella salvaguardia della vita familiare e personale dell'immigrato. Anche questo è un elemento che dava alle commissioni territoriali ampia capacità di poter intervenire, concedendo la protezione speciale. Nel frattempo che la protezione speciale, che prima veniva indirizzata su casi speciali, è diventata una specie di sanatoria per regolarizzare tutti quelli che si vedevano respinta la richiesta di diritto di asilo e di protezione sussidiaria

noi per superare il problema della clandestinità li trasformiamo tutti in regolari. Poi ci accusano che non riusciamo a rimpatriarli e ci credo: se hanno in mano un permesso di soggiorno. Hai voglia a rimpatriarli, Colleghi, naturalmente sapete che non si possono esporre cartelli. Cosa facciamo con il nostro emendamento? Riportiamo la protezione speciale nelle sue condizioni di specialità. Ma è evidente che gli obblighi internazionali e costituzionali sono garantiti. Se qualcuno rischia di essere perseguitato per orientamento religioso, politico, sessuale e identità di genere, volete che non gli venga concesso il permesso? Noi non abbiamo mai chiesto di togliere questo. Alla luce di questo, bisogna spiegare bene ai cittadini italiani e a tutti che la nostra proposta...

Abbiamo compreso benissimo e non mi costringente a richiamarvi nominalmente. *(Applausi)*. Presidente Romeo, un momento. Colleghi, sapete tutti benissimo che non si possono esporre cartelli, altrimenti gli assistenti verranno a ritirarli.

Il centrodestra legittimamente, a differenza di chi ha posizioni diverse, sostiene che preferisce e vuole regolarizzare dei casi specifici e giusti. Ci sono: c'è il decreto flussi, solo la protezione e il diritto d'asilo, c'è la protezione sussidiaria, c'è una forma di protezione speciale. Non possiamo però usare la protezione speciale sostanzialmente per dare in mano un permesso a tutti, dicendo che in questo modo si integrano, anche perché su 45.000 protezioni speciali ottenute solo 2.600 sono convertite in permessi di lavoro. Quindi, non è dando un pezzo di carta che automaticamente ci sono l'integrazione e il lavoro. Non è questo il punto, tant'è vero che nel decreto noi insistiamo affinché venga potenziata l'integrazione di coloro che hanno tutti i diritti a rimanere sul nostro territorio.

né più né meno a come era stata pensata - a nostro giudizio - dai decreti Salvini, ossia per casi speciali e non per tutti. *(Applausi)*. È legittimo. Questo è il succo dell'emendamento. un punto formale che viene tolto. Ci mancherebbe altro, c'è la discussione se metterlo o metterlo, meglio metterlo o non metterlo. Facciamo una cosa, Presidente: questi obblighi costituzionali e comunitari mettiamoli come postilla a tutte le leggi che facciamo. Se dobbiamo ribadirlo perché abbiamo paura che non li osserviamo, scriviamolo. A noi va bene comunque. *(Applausi)*.

il mio intervento non è teso a verificare quanta marcia indietro sta facendo la maggioranza su questo punto. Di marcia indietro si tratta e, siccome abbiamo tutti tanta esperienza qua dentro, lo abbiamo capito in modo molto chiaro. potremmo anche essere parzialmente soddisfatti di aver indotto, insieme probabilmente ad altre realtà istituzionali, questo parziale ripensamento, che non ci soddisfa, ma in qualche modo sentenzia il fatto che voi avete commesso un errore di valutazione, anche molto grossolano. Il punto è un altro: voi non lo potete fare in Aula *(Applausi)* e quest'Aula non può essere messa sotto schiaffo di iniziative che arrivano in corso d'opera. Per quale ragione non lo potete fare in Aula? La riformulazione di un emendamento in corso d'opera prevede compensazioni da parte degli altri soggetti titolari della discussione, e cioè eventuali subemendamenti. Presidente, mi rivolgo a lei, rivolgo a lei, che in questo momento ci deve dirigere: noi ovviamente prendiamo atto della volontà della maggioranza. Le chiederei di governare in maniera ordinata questa richiesta di modifica con una sospensione, affinché si riconvochi la Commissione,

minuti di sospensione per poter valutare la riformulazione ed esprimersi anche compiutamente sulle votazioni, li concederò, sapendo che non è possibile

Vorrei semplicemente sottolineare anch'io la situazione veramente grottesca nella quale ci troviamo. Per ricapitolare anche ai colleghi che non fanno parte della 1a Commissione, e che quindi non sanno esattamente cosa è accaduto in questi giorni,

capite bene che siamo in un autentico stato confusionale che, però, dobbiamo spiegare al Paese, perché altrimenti non si capisce a cosa è dovuto. È dovuto a una ragione evidente: a un conflitto tra le forze che compongono la maggioranza parlamentare.

a 10.000 ricorsi e a una situazione palesemente a rischio incostituzionalità. È stato richiamato ed è assolutamente evidente che è così. E probabilmente c'era poi all'interno della stessa maggioranza chi voleva invece in qualche modo utilizzare fino in fondo gli strumenti

Questa è la verità della vicenda. È chiaro che, se tu interpreti il ruolo di Governo, ma continui a fare esattamente quello che hai fatto negli anni... avete detto tutto e il contrario di tutto in questi giorni. Dinanzi all'obiezione di chi, come le forze di opposizione, tutte - devo dire - ha avanzato argomenti argomenti francamente anche molto ragionevoli, addirittura a un certo punto ci avete raccontato - pensate voi - che la protezione speciale non esiste in alcuna parte del mondo.

anche altri 18 ordinamenti europei hanno una legislazione come la nostra sul punto. Era quindi stata raccontata una bugia.

Come si può dire in quest'Aula, davvero impunemente, che il processo della protezione speciale serve a costruire una nuova sanatoria, a fermare l'invasione e tutte le stupidaggini che abbiamo ascoltato in questi giorni?

però basta propaganda. Se volete governare il Paese, avete preso i voti, siamo in democrazia, siete in maggioranza, fatelo senza ricorrere alla propaganda permanente che utilizzate come unico metro di governo.

È mio costume rispondere a delle domande che mi vengono fatte su un aspetto delicato che sta giustamente richiamando l'attenzione dell'Aula e, quindi, sull'emendamento in questione. Sono state dette delle cose non vere. Si fa propaganda? No: si fanno leggi. C'è chi fa ostruzionismo e chi vuole cambiare le leggi in base a un mandato che questa maggioranza ha avuto dal corpo elettorale *(Applausi)* e non perché uno si sveglia la mattina e vuole correggere le leggi. È una materia delicata e controversa? Sì: è una materia delicata e controversa. Non ci sono norme analoghe a quelle italiane in altri Paesi - e lo dico alla Presidenza, per non rivolgermi al senatore De Cristofaro - perché le fattispecie codificate in Italia non hanno uguali per la loro ampiezza, generosità e portata demagogica, che si sono stratificate nel corso degli anni. Poi ogni Paese ha le sue norme e le sue regole.

cambiano le regole della protezione speciale, ve lo dovete mettere bene in testa. Non facciamo propaganda, ma cambiamo l'ordinamento legislativo dello Stato. Potrei fare mille esempi. Con il testo, se mai sarà approvato, con il numero corretto che la Presidente giustamente citava prima, ad esempio

nel proprio Paese e non serve venire in Italia. Viene quindi cambiata profondamente la regolamentazione demagogica che è stata portata ad estreme conseguenze, per noi sbagliate, nel 2020. Siccome chi governava nel 2020 oggi è all'opposizione, abbiamo il diritto democratico di scrivere norme e lo stiamo facendo con questo emendamento *(Applausi)*, che cambia profondamente le regole. Potrei fare mille altri esempi in cui questa protezione speciale non ci sarà più. Non viene completamente abolita, e l'abbiamo sempre detto; personalmente, sono intervenuto in Parlamento, sui giornali e nei dibattiti pubblici e televisivi chiarendo che non viene abolita con questa normativa, ma viene rivista in senso più restrittivo. Dopodiché si tiene il dibattito parlamentare. C'è un punto controverso, il punto 1.1. 1.1. Se chi presenta un emendamento prende atto del dibattito, dovreste essere contenti della sua utilità su un punto della questione, e non dire che c'è confusione; la confusione non c'è. Il decreto-legge è stato fatto e viene migliorato; voi avete fatto ostruzionismo, mentre noi facciamo leggi per lo Stato, per dare maggiore sicurezza sui temi

C'è un punto controverso? Per noi non è decisivo. C'è un riferimento ad accordi internazionali? Che restino pure. Ma tutto il resto, che modifica in maniera sostanziale la protezione protezione speciale, resta se l'emendamento verrà approvato. C'è la serietà dell'ascolto: noi in Parlamento ci stiamo per confrontarci, non per fare soltanto crociate polemiche e lanciare insulti. Quindi, se ascoltiamo, riflettiamo e miglioriamo le norme, lo facciamo perché siamo parlamentari seri,

evidentemente il presidente Romeo non è stato in grado, nonostante la passione che ci ha messo, di spiegare all'Assemblea le caratteristiche che in qualche modo sottintendevano i contributi del senatore Gasparri, rispetto ad alcuni limiti che questo quadro normativo così confuso ha in merito al contesto internazionale. La cosa che vorremmo dirle a nome di tutto il Partito Democratico, Presidente, dieci minuti anziché cinque per far sì che il sottosegretario Molteni capisca meglio la riformulazione del senatore Gasparri, noi ci siamo e ovviamente siamo disponibili a continuare per tutta la sera, pur di completare il lavoro emendativo,

Signor Presidente, sono a chiedere, per il suo tramite, l'intervento illustre del Presidente della Commissione bilancio a tutela del fatto che questa riformulazione non abbia profili finanziari.

dai propri familiari perché volevano che sposasse un uomo nel proprio Paese, un caso di matrimonio forzato. Ebbene, Saman è stata uccisa perché tornò a casa per prendere i documenti che le servivano per poter svolgere una vita normale nel nostro Paese, tra cui anche il permesso di soggiorno. Per questo già nella scorsa legislatura tutto il Parlamento si attivò - devo dire sotto l'impulso soprattutto del MoVimento 5 Stelle e della collega deputata Stefania Ascari - per esaminare una legge che tutelasse le donne vittime di questo reato e consentisse loro di avere immediatamente il permesso di soggiorno. Quell'*iter* si interruppe con il cadere della legislatura.

fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento. Devo dire che, avendo illustrato questo emendamento, avevo anche trovato una certa sensibilità e una propensione all'accoglimento da parte del Governo e della maggioranza e ho ricevuto anche una telefonata da parte della segreteria della ministra Roccella che mi garantiva che avrebbe fatto ulteriori approfondimenti, perché naturalmente nel merito erano d'accordo. Devo dire che con grande sconcerto grande sconcerto rileviamo l'assoluta scorrettezza del senatore Gasparri nell'aver voluto inserire questo accorgimento e questa misura in un emendamento per noi dell'opposizione assolutamente invotabile, perché è l'emendamento sul quale si è discusso tutta l'ultima ora, che sostanzialmente elimina o svuota di significato la protezione speciale. Trovo che questo sia un comportamento politicamente davvero molto scorretto, che va anche contro l'atteggiamento che il Governo, nella persona del sottosegretario Molteni, aveva tenuto in Commissione e che abbiamo apprezzato. Chiedo quindi quantomeno che venga data alle forze di opposizione, che sono state promotrici di questa iniziativa, in realtà il MoVimento 5 Stelle in particolare, la possibilità di votare a favore di questa iniziativa, ossia quella del contrasto al matrimonio forzato e di concedere il permesso di soggiorno alle vittime di tale reato, e quindi di votare per parti separate questo emendamento, in particolare il comma b) della prima parte, che reca proprio la norma che prevede questo accorgimento a tutela delle donne, delle ragazze e delle bambine vittime di questo reato.

abbiamo apprezzato lo sforzo che questa maggioranza ha cercato di fare, con la rivisitazione del tema della protezione speciale.

perché si era detto che, se approvato questo emendamento, sarebbe stato ritenuto assorbito il seguente, senatrice Maiorino, che ha il medesimo contenuto di quella parte dell'articolo a cui faceva riferimento la senatrice Maiorino. Poiché sull'emendamento 7.0.1 c'era un parere ostativo della 5a Commissione, prima di mettere in votazione l'emendamento

De Cristofaro e da altri

Ho memoria di cose bellissime e qualcuna di molto triste. Ricordo di una persona dolcissima, competentissima e un po' eroica, che si chiamava Andreatta. In una sera come questa, ed era presidente Violante, mi permisi di dire che l'"accanimento" di troppe votazioni impreviste metteva, non dico a repentaglio - purtroppo è accaduto la vita delle persone. Non voglio drammatizzare, signor Presidente, ma quando l'orario si protrae in maniera imprevista è in qualche modo imprevedibile, perché la necessità e l'urgenza sono relative. Nonostante l'importanza enorme del provvedimento, spesso criticato in maniera un po' fantasmagorica, esiste lo *stress*. Su questo non mi maschero. Nonostante sia definito fragile, direi che la "metto nei fondelli" a parecchie persone: sono forte abbastanza. Forte non a livello di prevaricare, ma di condurre le nostre battaglie. Esistono però persone che, non prevedendo, hanno magari da fare terapie che non vogliono esplicitare,

mette a rischio, certo moderato - ma è successo con Andreatta e non solo - la vita delle persone. Mi permetto di dire intanto se la necessità e l'urgenza sono tali - forse come in questo caso, lo dovrebbero prevedere il mio Capogruppo o i nostri Presidenti di Commissione

non mangiare a una certa ora non è un problema di fame, ma va previsto, altrimenti davvero - io scateno magari in maniera un po' volgare il principio di precauzione - condurre costantemente in questo modo - non certo per colpa sua, anzi complimenti per la

di sospendere quanto prima i lavori per evitare magari che si inciampi per terra, che ci prenda ci prenda una crisi depressiva, perché spero che non accada più quello che è accaduto al grande - e non solo grosso - Andreatta.

questo è compatibile, andiamo avanti;

Mi stanno rendendo edotta su una modifica in corso d'opera su alcuni punti che avevamo già in programma domani, per cui sto cercando di capire cosa significa questo, in modo da poter concordare come proseguire.

Signor Presidente, io concordo totalmente con quanto detto dal senatore Malan. Domani, anche grazie alla comunicazione che lei ci ha dato, abbiamo un ordine del giorno ridotto, per cui possiamo tranquillamente iniziare il lavoro alle ore 10, ripartendo dall'articolo che abbiamo lasciato. Peraltro mi faccia dire che il senatore Guidi ha posto una questione importante: quando ci assumiamo la responsabilità di chiudere una seduta entro un determinato orario, è vero che ci possono essere degli imprevisti, ma dobbiamo considerare anche tutta una serie di questioni che magari per alcune persone sono rilevanti

non penso - lo dico al senatore Malan e gli altri colleghi - che possa metterci in difficoltà se iniziamo mezz'ora prima: o ci diamo la garanzia comune o ci diamo la garanzia comune che l'esame delle mozioni finisce prima del *question time;* altrimenti è evidente che rischiamo che si metta in discussione l'esame e la votazione delle mozioni.

Presidenti dei Gruppi parlamentari. Per quanto mi riguarda, se fate una valutazione per cui si inizia alle ore 9,30 e finiamo in tempo, va bene; se iniziamo alle ore 10, noi dobbiamo avere la certezza che le mozioni vengano votate prima del *question time.*

l'*iter* della mozione non è proprio rapidissimo, perché prevede comunque una discussione generale e delle dichiarazioni di voto. Dobbiamo anche considerare le dichiarazioni di voto su questo decreto-legge. Quindi, sono tre ore solo per le dichiarazioni di voto,

Presidente, anche per noi va benissimo la proposta del senatore Malan di iniziare domani mattina alle ore 10. Ricordo al senatore Boccia che avevamo già stabilito in Conferenza dei Capigruppo di la mozione e poi con il *question time*. Siccome siamo persone per bene e rispettiamo gli accordi, faremo esattamente quello che abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi)*. Signor Presidente, per il nostro Gruppo l'orario di inizio di domani non è determinante, ma è determinante che si possa, prima del *question time*, discutere la mozione che è calendarizzata. Con questa garanzia, noi possiamo iniziare anche alle ore 10, ma ci deve essere la garanzia

solo per dare la garanzia sulle mozioni: se dovessimo essere in ritardo, vorrà dire che rinunceremo all'intervento o faremo solo cinque minuti di dichiarazione di voto per consentire il voto della mozione.